L'ordine del giorno reca la discussione congiunta della Risoluzione della 3a Commissione permanente sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie» (COM (2008)

la relazione che a suo tempo presentai alla Commissione esteri e da cui è derivato il documento al nostro esame mi consente di concentrare l'attenzione su due essenziali argomenti:

Naturalmente, ribadisco i contenuti della mia relazione e specialmente quelli della risoluzione conclusiva, che avendo sapientemente raccolto l'essenza di un vasto dibattito fu approvata all'unanimità. Oggi colgo, nelle mozioni presentate, punti significativi di convergenza, ma anche diversità di analisi e di proposta che, nonostante tutto, spero possano ricomporsi nuovamente in una sintesi unitaria. L'immigrazione clandestina l'immigrazione in generale condizionano il nostro presente e incideranno ancora di più sul nostro futuro. È questione troppo importante per lasciarla in balìa delle ordinarie contese politiche. Vorrei innanzitutto insistere sulla necessità di contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina. Essa costituisce la patologia di un fenomeno largamente positivo, perché aggrava l'andamento della delittuosità complessiva, suscita allarme sociale e rende più difficile la stessa integrazione degli immigrati regolari. Non a caso, la lotta ai clandestini ha contrassegnato lungamente la politica europea sull'immigrazione. però, l'opinione prevalente in Europa - e cito documenti ufficiali - è che una gestione strutturata della migrazione legale ed una efficace lotta contro l'immigrazione clandestina vadano considerati anche come strumenti per favorire le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo. In altri termini, il mezzo più efficace contro l'immigrazione clandestina è il governo intelligente dell'immigrazione regolare, ed entrambe devono essere trasformate in forze positive a favore dello sviluppo. Sappiamo tutti, onorevoli colleghi, che ormai da diversi anni l'Italia ha bisogno dell'immigrazione per mantenere il tasso attuale di popolazione attiva e il corrispondente livello di sviluppo. Certamente, il nostro futuro benessere dipenderà dalla nostra capacità di attrarre e integrare lavoratori stranieri. Sbaglieremmo, tuttavia, se considerassimo l'immigrazione soltanto come una necessità, perché la mobilità umana è il tratto più saliente della globalizzazione ed il segno di un'ampia curvatura della storia, che dobbiamo percorrere con avvedutezza se non vogliamo uscire fuori strada. Le dimensioni del fenomeno sono note e tendono a crescere. Un sondaggio recente, condotto dalla *Gallup* in 135 Paesi diversi, rivela che ben 700 milioni di persone in età adulta lascerebbero definitivamente il loro Paese se appena ne avessero la possibilità. Prima o poi partiranno, sospinti dalla forza incontenibile degli squilibri economici, demografici e politici che affliggono il nostro pianeta. La prima grande ondata migratoria ci ha colti quasi alla sprovvista, mettendo a nudo tutta la nostra inadeguatezza, ma anche lasciandoci intravedere le strutture e gli strumenti giuridici e culturali dei quali abbiamo bisogno per governare l'accoglienza e l'inserimento dei migranti nel nostro tessuto economico e sociale. Non possiamo farci prendere alla sprovvista una seconda volta, né tanto meno possiamo arroccarci nella cieca difesa dell'identità minacciata alimentando la paura della diversità specialmente presso i gruppi sociali economicamente e culturalmente più deboli. Quello che oggi ci chiede l'approccio globale all'immigrazione non è la resa delle nostre identità, bensì l'apertura delle nostre società ad energie umane e culture diverse che possono arricchirle e farle progredire. Personalmente sono convinto che le radici giudaico-cristiane hanno una grande e vitale forza unitiva, di cui deve nutrirsi la costruzione europea. Ma l'unità dell'Europa non può basarsi esclusivamente sul passato, cioè soltanto sulle tradizioni e sulle culture nazionali che ancor oggi per tanti aspetti ci dividono. Deve basarsi invece su un progetto comune per il futuro, un progetto che ci unisca veramente. Questo futuro comune lo possiamo offrire alle minoranze in crescita degli immigrati mediante una gestione oculata ed umana dei processi migratori. Chiedo a me stesso, onorevoli colleghi, ed a quelli di voi che hanno interesse all'argomento: se per oltre 2000 anni le nostre società sono cresciute sull'antico ceppo greco-romano e giudaico- cristiano, perché mai non dovrebbero continuare a crescere con l'apporto di altre sensibilità ed altre culture, come fanno ancora oggi, attraverso l'immigrazione, gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda? Che senso ha coltivare l'incubo di Babele, confusa tra molte lingue e poi atterrata, mentre a New York e nelle nuovissime capitali del Golfo Persico si parlano 150 lingue diverse? Certo, la storia e le identità pesano, ma la storia avanza e le identità si evolvono, e si evolvono aprendosi,

E allora non possiamo fondare la cittadinanza sull'etnia cristallizzata e neppure sulla religione,

dice Giuliano Amato -manca di universalismo. E proprio per questo - aggiungo io - è assai distante da quella visione da quella visione cristiana che taluni sembrano avere acquisito in esclusiva. Certo, non è facile impostare e realizzare una politica per l'immigrazione all'altezza dei tempi che vengono. L'Unione europea ha poche risorse, come ben sa il ministro Maroni; tuttavia riesce a produrre idee che sono capaci di armonizzare i programmi dei singoli Governi. Pertanto, un'accorta politica italiana deve oggi fare prevalente affidamento sulle risorse proprio ed allo stesso tempo deve puntare sull'orizzonte europeo, allungando lo sguardo all'obiettivo lontano ma non impossibile di un governo mondiale dell'emigrazione. Oggi i Governi dei maggiori Paesi europei sono costretti, come il nostro Governo, a procedere tra Scilla e Cariddi: mentre da un lato debbono garantire i flussi richiesti dal mondo economico, dall'altro debbono tranquillizzare le loro opinioni pubbliche in apprensione per la sovranità, l'identità e la sicurezza. Tra questi due scogli deve passare la nostra esigenza di fondo, quella cioè di inserire proficuamente migliaia e migliaia di lavoratori stranieri e i loro familiari nel nostro tessuto economico e sociale, garantendo almeno la pacifica convivenza di identità diverse nel rispetto rigoroso dei nostri ordinamenti e delle nostre leggi. Le difficoltà sono enormi, come attestano sia le manifestazioni di intolleranza, xenofobia e razzismo da parte dei nostri connazionali, sia le reazioni organizzate e in taluni casi violente da parte degli immigrati; reazioni cui si sono aggiunti, più di recente, sanguinosi scontri interetnici e guerriglia urbana. Da Rosarno a via Padova giungono segnali che non possiamo sottovalutare; infatti, con la crisi in atto e con l'accentuarsi del disagio sociale c'è da temere il peggio. Il rischio maggiore viene dagli immigrati di seconda generazione, spesso emarginati e delusi, i quali in questo contesto possono formare massa critica e scatenare protesta e violenze; è dunque innanzitutto su di loro che dobbiamo intervenire, sottraendoli all'emarginazione e confidando sulla loro naturale attitudine a conciliare la modernità con la cultura dei padri. In Italia si è fin troppo discusso di integrazione alla maniera francese, inglese, olandese o portoghese: alla maniera cioè di Paesi che hanno preso dimestichezza con l'immigrazione molto prima di noi, sulla scia della loro esperienza colonialista. Ma al di là di certe astrazioni, in realtà non esistono modelli compiuti e ben riusciti che si possano tranquillamente acquisire; esistono invece pratiche efficienti di gestione pubblica dell'immigrazione, che dobbiamo studiare ed adattare alla realtà italiana. Altre dobbiamo inventarle. Occorre pertanto un progetto nazionale per l'immigrazione, che definisca la nostra capacità complessiva di accoglienza sia in base alla forza lavoro che vogliamo attirare, sia in base ai servizi sociali e agli strumenti di integrazione che possiamo offrire. In tale progetto debbono trovare armonica composizione le questioni più controverse evocate dalle mozioni presentate. Mi riferisco alla disciplina dell'asilo, dei respingimenti individuali alla frontiera e del rimpatrio, alla durata dei visti e allo sfruttamento del lavoro nero, al dialogo interreligioso, al diritto di voto nelle elezioni amministrative e alla cittadinanza. Più in generale, come ha giustamente sostenuto il ministro Maroni in una recente intervista, c'è bisogno di un cambio di passo nelle politiche attive per l'integrazione: c'è bisogno cioè di puntare decisamente sulla ricostruzione del modello sociale, mobilitando i poteri locali e regionali insieme alle risorse impareggiabili del volontariato italiano. L'anima di un tale progetto non può che essere la scelta del pluralismo, in virtù del quale più religioni e più culture possono convivere e arricchirsi reciprocamente nello spazio umano e politico della società aperta e della nazione europea, evitando allo stesso tempo il caos multietnico e il grigiore del sincretismo. Ciò che importa è che gli immigrati, una volta stabilizzati in Italia, entrino a far parte della storia italiana e contribuiscano a fabbricarla con un comune senso dei diritti e dei doveri. Facile a dirsi, difficile a farsi; molti Paesi, seppure in contesti diversi, però lo hanno già fatto e continuano a farlo tessendo ogni giorno la tela faticosa dell'integrazione. L'integrazione non è una pratica, una procedura umanitaria, ma una gigantesca operazione politica che sfida la lungimiranza della società civile e delle istituzioni, perché le chiama a costruire qualcosa di veramente nuovo dopo tre secoli dominati dalla cultura e dalle vecchie chiusure degli Stati nazionali. Questa impresa, onorevoli colleghi, è affidata anche a noi. Penso che riusciremo ad avviarla bene se sapremo alzare lo sguardo al di sopra delle divisioni e dei reciproci sospetti che finora hanno bloccato il confronto politico sul tema davvero epocale dell'immigrazione.

della Commissione affari esteri sui problemi legati all'immigrazione con quello sulla mozione da noi presentata con riferimento alla corretta interpretazione da parte dello Stato italiano della disciplina in materia di tutela del diritto di asilo e di protezione umanitaria ci impone, ancorché nella brevità dei tempi che ci sono stati concessi rispetto ad un tema estremamente complesso e importante, di intervenire su entrambe le questioni. Per ragioni di brevità, cercherò di fare solo alcune considerazioni di natura sintetica, partendo dal presupposto che sottoscrivo dalla prima all'ultima parola la relazione che il senatore Pisanu ha svolto in quest'Aula e anticipo che voteremo la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione affari

ma perché nel merito credo che l'approccio che la Commissione affari esteri ha dato, all'unanimità, al tema dell'immigrazione, anche rispetto all'esatta individuazione delle responsabilità e delle competenze (in parte eluse e in parte non sollecitate) che l'Unione europea ha su questo tema, collochi esattamente lo scenario della frontiera dell'immigrazione e del ruolo che l'Italia deve avere nell'ambito delle sue competenze, senza rincorrere il facile alibi di scaricare sull'Europa le inadempienze o le inefficienze che vi sono obiettivamente nel contrasto all'immigrazione clandestina e nella gestione dei flussi: quella che il presidente Pisanu ha definito la gestione intelligente dell'immigrazione regolare. Sono

e sul tema della tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come il diritto di asilo, e che devono trovare soluzione in una disciplina omogenea e unitaria. Si tratta di una disciplina che, da un lato, proprio per la complessità del fenomeno

di recepirla a proprio piacimento, creando di fatto una legislazione diversificata che vulnera la possibilità di una politica unitaria in tema di immigrazione, di integrazione e di contrasto all'immigrazione clandestina. della normativa di principio che è contenuta nelle direttive comunitarie, la disciplina di dettaglio che ciascuno Stato membro prevede è sostanzialmente diversa da uno Stato rispetto ad un altro, ciò finisce per un'altalenante forma di migrazione interna o di immigrazione interna agli Stati dell'Unione, una concorrenza diversa all'interno degli Stati dell'Unione che non agevola il percorso né di integrazione, né di gestione intelligente dei flussi, ma che è funzionale solo a creare ulteriori a creare ulteriori elementi di disagio, di conflitto e di disintegrazione. Per ragioni di brevità, su questi aspetti non mi soffermerò, perché essi sono stati oggetto di una puntuale ricognizione che hanno fatto il presidente Pisanu come relatore e la Commissione nell'approvare questa risoluzione. Voglio però sottolineare alcuni altri aspetti. È evidente, come diceva il senatore Pisanu nel suo intervento, che sull'immigrazione qualunque approccio che sia di natura ideologica

qual è la mutevolezza del fenomeno migratorio. Rispetto a questo, credo che non si possa immaginare, come fino ad oggi si è fatto, una politica dell'immigrazione statale che sia solo circoscritta alla individuazione di misure sanzionatorie che però

sul reato di immigrazione clandestina che peraltro stenta a decollare, perché non fa altro che intasare i tribunali; possiamo scrivere tutto ciò che vogliamo, ma se poi a queste norme non si riesce a dare pratica attuazione perché ciò è obiettivamente impossibile, abbiamo sostanzialmente prodotto due risultati negativi: il primo è che il principio di legalità non viene garantito nella sua effettività; il secondo è che immaginiamo di affidare solo al messaggio ideologico la soluzione di un problema, che invece ha necessariamente bisogno di tanti altri elementi che non sono solo quello dell'esibizione di una faccia feroce a cui poi non corrispondono i fatti concreti. Se non fosse così, dovremmo anche fare un'analisi dei dati. In questo Paese si sono susseguite tre regolarizzazioni: una regolarizzazione, o sanatoria che dir si voglia, fu fatta con riferimento alla legge Turco-Napolitano; una seconda, che ha certificato il fallimento della legge Turco-Napolitano, fu fatta dal governo Berlusconi e portò alla emersione

questo fenomeno così diffuso di irregolarità, e altrettanto dobbiamo dire con onestà, se vogliamo evitare di fare della facile demagogia dell'ultima regolarizzazione parziale che è stata proposta dai Gruppi di opposizione e che ha trovato accoglimento solo per una parte, cioè per la regolarizzazione di colf e badanti, e che ha fatto emergere anche l'inefficacia degli strumenti della legge Bossi-Fini, che comunque hanno confermato quel circuito dell'irregolarità che tutti, a parole, vogliamo contrastare. Allora, è evidente che non basta solo immaginare di intervenire sul settore della repressione (cosa estremamente importante), ma dobbiamo anche porci il problema di capire se le regole che noi abbiamo introdotto con riferimento al mercato del lavoro extracomunitario (e quindi con riguardo all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro extracomunitario) siano efficienti, oppure se non contribuiscano in qualche modo a determinare la situazione

i clandestini che sono ristretti nelle carceri italiane (che sono circa il 30 per cento della popolazione carceraria) dovevano essere espulsi, non capisco come mai, a distanza di un anno dall'entrata in vigore di quella disciplina, il dato percentuale

abbiamo introdotto un secondo tema, che è quello che riguarda la mozione sui rifugiati. Dobbiamo infatti avere chiaro un principio, altrimenti rischiamo di

dei soggetti che sono rifugiati o richiedenti asilo deve essere sempre e comunque rispettato. È un principio che va rispettato ogni qualvolta lo Stato italiano, indipendentemente dalla territorialità della sua posizione, ha giurisdizione su questa materia.

Ad ogni modo, al di là di questo (che potrebbe essere oggetto di facile polemica), andiamo a verificare se la Libia, a cui abbiamo delegato un compito che comunque attiene al rispetto delle norme costituzionali del nostro Paese, gestisce concretamente oppure no questo principio secondo

(perché nessuno è nelle condizioni di fare degli accessi nei campi libici per verificare se sono rispettate queste condizioni), uno Stato e un Parlamento responsabili devono assumersi la responsabilità di affrontare questo tema se vogliono realmente operare e distinguere tra il contrasto all'immigrazione irregolare

Signor Presidente, colleghe e colleghi del Senato, signori del Governo, nell'ultimo mezzo secolo i processi di sviluppo hanno stretto i legami economici e sociali tra Paesi e continenti, posto in contatto società un tempo estranee e lontane, accorciato le distanze fisiche ed accresciuto la mobilità delle persone e delle forze di lavoro. Lo sviluppo però, pur elevando i livelli di vita in gran parte del mondo, non ha attenuato le disuguaglianze tra Paesi, anzi, in vaste regioni, ha approfondito il divario economico tra Paesi ricchi e Paesi poveri e, quindi, l'incentivo dei secondi a migrare verso i primi. D'altro lato, i processi demografici stanno provocando - in vaste aree del mondo sviluppato - un ristagno o un declino della popolazione giovane e adulta ed un'intensa domanda di lavoro immigrato proveniente da Paesi nei quali la dinamica demografica è ancora molto vivace. Questi processi accrescono le spinte ai movimenti internazionali di lavoratori e di famiglie, che però avvengono in un pericoloso vuoto di regole condivise, particolarmente grave perché gli interessi dei Paesi di origine sono in contrasto con quelli dei Paesi di destinazione e perché le aspettative e le aspirazioni dei migranti non trovano né rappresentanza, né protezione. Sintomatico il fatto che le convenzioni internazionali concernenti i diritti dei migranti e delle loro famiglie cadano nel disinteresse degli Stati, che non esista un embrione di governo globale delle migrazioni potente Organizzazione mondiale del commercio), che quasi tutti gli Stati rifiutino di assegnare anche una minima quota della loro sovranità nazionale in tema di migrazioni ad organismi sopranazionali. Questo vuoto di governo sottrae valore al contributo positivo che le migrazioni possono dare, e in effetti danno, ai processi di sviluppo dei Paesi di partenza e di quelli di arrivo, ed alla crescita dei livelli di vita dei migranti. Nel quadro internazionale sinteticamente descritto, nei Paesi del Nord del mondo sta facendosi strada molto lentamente - troppo lentamente vorrei dire - la convinzione che le politiche migratorie debbano imboccare un nuovo corso, che debbano diventare una parte integrante della politica estera degli Stati, che debbano assumere una posizione centrale nelle politiche di cooperazione allo sviluppo, contemperando gli interessi dei Paesi di origine - spesso colpiti dal depauperamento del loro capitale umano con quelli dei Paesi di arrivo e con quelli dei migranti stessi, garantendone e proteggendone i diritti fondamentali. Queste convinzioni debbono rapidamente convertirsi in azioni concrete ed a questo nuovo corso è particolarmente interessato il perché l'Italia, nella geografia delle migrazioni internazionali, occupa un'area strategica quanto delicata. Tra i grandi Paesi europei è quello demograficamente più debole per la bassissima natalità, solo in parte frazionale moderata dalla più alta (ma non altissima) natalità della componente straniera; per il rapido assottigliarsi della popolazione giovane e il velocissimo aumento di quella anziana e molto anziana. Tra i grandi Paesi europei è stata meta di flussi migratori tra i più intensi, Tra i grandi Paesi europei è quello geograficamente più prossimo al continente africano ed alle spinte migratorie provenienti dal Sud del mondo. Tra i grandi Paesi europei - assieme alla Spagna - esprime una domanda di lavoro spesso disattesa dalla insufficiente offerta autoctona: la esprime per la modestia del *welfare* familiare, che aumenta la necessità di lavoro straniero in aiuto delle famiglie, e per l'estensione di settori ad alta intensità di manodopera. Diamo un'occhiata alle statistiche per convincersi dell'eccezionalità del caso italiano: nel 2009, a fronte di 570.000 bambini con meno di un anno

Un'Italia senza migrazioni sarebbe un Paese più piccolo, meno dinamico e competitivo, con maggiori squilibri tra generazioni e più lento sviluppo. Sono, queste, alcune delle ragioni (quelle più evidenti)

ma fenomeni strutturali; aggiungo: destinati a durare in forma intensa per qualche decennio - una volta superata la grande crisi economica in corso - e ciò anche nel caso di una consistente ripresa demografica, della quale, peraltro, non si rilevano avvisaglie Occorre perciò che le politiche prendano atto di questa situazione ed impostino la propria azione in conseguenza. Per esempio, occorre non confidare nell'illusoria convinzione che la migrazione di breve periodo possa soddisfare le necessità migratorie del Paese. Le esperienze storiche di Paesi che hanno puntato su un'immigrazione di brevissimo o breve periodo (per esempio, la politica del "lavoratore ospite" in Germania), nell'intento di minimizzare il radicamento e l'investimento in integrazione, hanno frustrato le aspettative dei legislatori. Infatti, la convergenza di interessi tra migranti, datori di lavoro e settori della società ha portato alla stabilizzazione di chi arrivava per soggiorni temporanei. una parte considerevole dei migranti desiderano insediarsi stabilmente nel Paese ospite e per loro vanno disegnate politiche a queste funzionali, tenendo conto che l'immigrazione che stabilmente si integra è anche quella che più concorre ad uno sviluppo stabile. mi onoro di essere il primo firmatario, impegna il Governo attuale a porre la migrazione in un quadro strategico più ampio, che non sia dominato esclusivamente dalle esigenze securitarie (alcune fondate, molte pretestuose). Con riguardo alla unanime risoluzione della Commissione esteri sull'atto comunitario «Rafforzare l'approccio globale in materia d'immigrazione» - sulla quale ha così bene riferito il presidente Pisanu concordiamo con l'imperativo di estendere il governo delle migrazioni bene al di là del contrasto - pur imprescindibile - all'immigrazione irregolare collocandolo - cito testualmente dalla risoluzione - «in una visione complessiva delle politiche di accoglienza e di asilo, della cooperazione allo sviluppo e della gestione dei rapporti con i Paesi di origine e di transito dei migranti». Approccio globale significa anche cooperazione, che va di nuovo dotata di quei mezzi e di quelle capacità drammaticamente venute meno negli ultimi due anni, a dispetto delle intese e degli accordi sottoscritti in campo internazionale. Sull'irregolarità la posizione del Partito Democratico è univoca, dall'epoca dell'approvazione della legge Turco-Napolitano. Essa va contrastata con fermezza ed efficienza, ma anche con saggezza. Una stima dell'ISMU con riferimento al 2007 ne valutava il numero, in Italia, in 700.000, cifra dalla quale vanno dedotte le quasi 300.000 regolarizzazioni di badanti e colf ma alla quale va aggiunto un numero imprecisato di nuovi ingressi nella situazione di irregolarità (soprattutto nuovi *overstayers*, anche per il blocco di nuove ammissioni legali) e i numerosi "nuovi" irregolari, divenuti tali per la perdita del lavoro e del permesso di soggiorno. L'alto livello di irregolarità è imputabile soprattutto a tre fattori che coerenti politiche potrebbero depotenziare: in primo luogo l'evasione, l'economia sommersa ed il lavoro nero. Più ampia è l'economia sommersa, più alta è la domanda di lavoro irregolare e maggiore è la domanda di irregolari stranieri. Ogni rallentamento o inversione di marcia nella lotta all'economia sommersa è uno stimolo oggettivo all'irregolarità. In secondo luogo, la normativa per l'assunzione legale di uno straniero (mediante la cosiddetta chiamata nominativa o numerica di uno straniero sconosciuto residente all'estero) è impervia, in particolar modo per famiglie, artigiani o piccoli imprenditori che spesso optano per l'assunzione (al nero) di un irregolare, regolarmente entrato, ma con visto scaduto. Infine, vi è la combinazione della brevità dei permessi di soggiorno, della macchinosità del loro rinnovo e del loro costo (sia quello monetario, diretto, sia quello indiretto) che rende alta la probabilità che un regolare diventi irregolare suo malgrado. La nostra mozione ravvisa nei tre fattori sopra riassunti il motore che alimenta l'irregolarità, che può essere frenata sia da coerenti politiche anti-evasione e pro-emersione, sia da sostanziali modifiche del regime normativo dell'immigrazione. Ciò può farsi introducendo - e sperimentandole, con l'introduzione di tetti numerici - nuove forme di ingresso legale più adatte a gestire un sistema migratorio complesso: ad esempio, la concessione di visti per ricerca di lavoro, con garanzie finanziarie o di *sponsor* istituzionali certificati, o la trasformazione, a determinate condizioni, del permesso di soggiorno breve in permesso per ricerca di lavoro. Inoltre, un Paese che ospita milioni di immigrati deve investire sulla macchina burocratico-amministrativa preposta al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, oggi clamorosamente lenta ed inefficiente. fine di evitare il succedersi di sanatorie e regolarizzazioni di massa, come quella dello scorso autunno, vanno introdotte forme di regolarizzazioni *ad personam* per coloro che contribuiscono all'emersione di fattispecie criminose legate all'immigrazione; per coloro che compiono atti di rilevanza umanitaria e sociale;

consentendo e incentivando il rimpatrio volontario degli irregolari, oggi paradossalmente precluso dalla normativa del pacchetto sicurezza. Il ministro Maroni sa bene che questo è un problema che va risolto. Signor Presidente, sull'immigrazione - e sui temi dell'integrazione, dei diritti politici e della cittadinanza degli immigrati che per brevità non posso affrontare - si gioca una parte rilevante del futuro del nostro Paese. Allargando lo sguardo alle dimensioni mondiali delle migrazioni potremo meglio capire ciò che sta avvenendo in casa nostra e - nel contempo - saremo indotti a dare un respiro largo alle politiche migratorie, a superare la logica esclusivamente securitaria, a valorizzare i diritti dei migranti, a non tradire le aspettative dei concittadini in una coesistenza serena con gli immigrati, a non agitare, suscitare o ingrandire paure non giustificate.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, illustrerò questa mozione come senatore della Repubblica, ma anche - se mi è consentito - come sindaco di un Comune della provincia bresciana, una provincia che purtroppo conosce il fenomeno dell'immigrazione.

di una provincia che è sempre stata accogliente e di un popolo disposto ad accogliere chiunque, ma che oggi inizia a manifestare segni

Quindi, non abbiamo una dimensione policentrica, come hanno altri Paesi, di comunità straniere sparse sul territorio nessuna delle quali prevalente. Noi - ripeto - abbiamo una forte presenza dell'immigrazione che viene dall'Est europeo

le attività che ti consentono di fare soldi in poco tempo sono lo spaccio di droga, lo sfruttamento della prostituzione o, peggio ancora, diventare manovolanza della criminalità organizzata. Bisogna distinguere all'interno di quel fenomeno che chiamiamo indistintamente immigrazione almeno queste due componenti, che sono completamente differenti.

Noi diciamo che, anche se sta commettendo reati di non particolare gravità, sta venendo meno a un patto di integrazione che deve stipulare con la comunità statale e con quelle locali che lo ospitano. Questo istituto dell'accordo di integrazione funziona bene nei Paesi che lo hanno già sviluppato.

Nella mozione n. 246 richiamiamo il famoso Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo dell'ottobre 2008, che spesso viene dimenticato, e che contiene cinque impegni molto chiari. Il primo impegno è di organizzare l'immigrazione regolare tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità di accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l'integrazione.

Dobbiamo pertanto seriamente valutare la nostra capacità di accoglienza tenendo conto della situazione economica che viviamo oggi. In questo Paese c'è una situazione di crisi drammatica.

in particolare, il ritorno nel loro Paese di origine degli stranieri in posizione irregolare. Il verbo usato in questo Patto europeo dovrebbe dirvi qualcosa: si parla di combattere l'immigrazione clandestina perché l'Unione europea capisce che siamo di fronte ad una situazione grave che va combattuta fino in fondo. I clandestini vanno rimandati nei loro Paesi di origine senza sconti, senza se e senza ma. Questo ci chiede l'Unione europea e così abbiamo fatto. Quando abbiamo introdotto il reato di clandestinità abbiamo semplicemente dato attuazione ad un impegno fondamentale del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo.

Il reato di clandestinità non nasce nel congresso di Fiuggi del 1995: sta in un disegno di legge dei ministri Andreotti, Scalfaro e Martinazzoli del 1986. Già allora era chiaro che bisognava far capire che chi entra in questo Paese violando le norme sull'ingresso e sul soggiorno non può essere tollerato in questo Paese; va rispedito nel suo Paese, perché viola il principale elemento di uno Stato che è la sua sovranità territoriale.

poi di creare un partenariato globale con i Paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le immigrazioni e lo sviluppo. In termini semplici,

del lavoro. Chiediamo che ci sia una costante correlazione fra l'immigrazione e il lavoro e che la crescita della presenza straniera sia legata alle effettive esigenze del mercato del lavoro. Dunque, non siamo favorevoli a sanatorie generalizzate

Credo che anche questo aspetto meriti una riflessione. Non possiamo continuare ad accogliere immigrati quando registriamo una disoccupazione interna di questa gravità. Per queste ragioni chiediamo al ministro Maroni di continuare nelle sue politiche sull'immigrazione e nella politica selettiva dell'immigrazione. Riceverà continue critiche, Ministro, ma lei continui nella sua opera!

il problema che oggi è posto all'attenzione del Senato è particolarmente critico perché si attaglia a questioni che afferiscono alla sfera sociale, antropologica e politica del nostro Paese. Nell'intervento dei miei colleghi e, in particolare, del senatore D'Alia sono stati usati termini quali «soggetti», «individui» per qualificare questo fenomeno e con riguardo agli stranieri. A me piace, invece, dire che questo è un problema che riguarda delle persone e non dei soggetti o degli individui. In Italia ci sono circa 3 milioni di cittadini stranieri in posizione regolare e circa 600-700.000 cittadini extracomunitari che sono entrati nel nostro Paese non attraverso le carrette del mare, ma attraverso

e un problema di integrazione nella sfera sociale del nostro Paese, che un Governo serio e una maggioranza come quella del PdL deve poter governare. Dietro al problema dell'integrazione di questi milioni di cittadini stranieri ci sono anche problemi di devianza, di intolleranza, ma anche di sfruttamento e di tratta degli esseri umani. Non è un segreto che ormai l'80 per cento dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti sia commesso da cittadini stranieri. non è un segreto che il 90 per cento degli omicidi delle donne nel nostro Paese è stato compiuto da cittadini stranieri ed, evidentemente, nel flusso dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione.

per far sì che la certezza del diritto potesse essere affermata anche in questo campo. Lo abbiamo fatto anche attraverso un aumento delle relazioni con i Paesi di provenienza di questi flussi migratori, in particolare, con quelli della sponda Sud del Mediterraneo. I dati

Non è un caso che questo principio si radichi non solo nella tradizione giudaico-cristiana, ma anche in quella previsione che Immanuel Kant teorizzò alcuni secoli fa: l'uomo prima di tutto e non l'uomo come fine. Non è un caso che le misure introdotte tengano presente che l'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo a tutti gli uomini, a tutti i cittadini e a tutte le persone che sono presenti nel nostro territorio, ma non sottrae gli stranieri allo Stato di diritto e all'obbligo di osservare le norme che questo Paese si è dato. Il rispetto della legalità e dello Stato di diritto è il principio fondamentale intorno a cui può ruotare una corretta politica dell'immigrazione: ciò significa rispetto della dignità umana, tutela e rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, ma anche riconoscimento dei doveri inderogabili che tutti i cittadini stranieri debbono osservare all'interno del nostro Paese. Il contratto d'integrazione per gli stranieri non è altro che tutto ciò.

il regime dei permessi di soggiorno siano commisurati al livello di legalità che deve essere garantito all'interno del nostro Paese. L'immigrazione è una risorsa, ma è anche un fattore di devianza. Non è un caso che metà della popolazione carceraria sia composta da cittadini extracomunitari. Noi intendiamo con questa mozione sostenere tutta la politica che il Governo ha fatto attraverso gli accordi bilaterali e di cooperazione con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Credo che sia un vanto il fatto che il Governo italiano, il presidente Berlusconi e il ministro Maroni abbiano concluso l'accordo con la Libia che ha impedito gli sbarchi e, quindi, lo sfruttamento e la tratta degli esseri umani, che invece avvenivano prima di questo accordo. Ecco quindi che le nostre mozioni impegnano il Governo a proseguire su questa strada, ma lo impegnano anche nelle sedi comunitarie a far sì che i Paesi dell'Unione europea dell'Unione europea possano accordarsi su questi temi e possano sostenere con maggior rigore e impegno il nostro Paese, che ha fatto della solidarietà e - se mi consentite - della carità e del sostegno ai Paesi più poveri un punto fondamentale della sua azione. Vorrei qui ricordare che il contributo finanziario dell'Italia alle agenzie umanitarie internazionali è, comunque, uno dei più alti al mondo. alti al mondo. La maggioranza vuole impegnare il Governo a rafforzare queste relazioni con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo appunto, un rafforzamento e un'attività diretta a corroborare le relazioni con i Paesi di flusso e di transito degli extracomunitari, attraverso una stretta vigilanza sulle politiche dei flussi, dei visti, dei permessi di soggiorno e delle regolarizzazioni, in modo tale che l'immigrazione possa costituire davvero, come detto poco fa dal senatore Pisanu, una risorsa capace di sostenere livelli di crescita e di reddito del nostro Paese ma, nel contempo, non possa determinare fratture con il sistema sociale e valoriale del nostro Paese che, lo ripeto, si radica nella tradizione greca, romana, e giudaico-cristiana. Sono valori imprescindibili, che pongono, sì, l'uomo al centro del sistema, ma impongono anche il rispetto delle norme e dei valori del nostro Paese. Chi viene in Italia deve sapere che troverà solidarietà e accoglienza, se si immetterà in un circuito criminale e violerà le regole che questo Paese si è dato, di fronte a lui troverà la maggioranza, il Governo e la legge a fronteggiare questi comportamenti. Conclusivamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la maggioranza auspica che il Governo rafforzi questa politica di governo dell'immigrazione che ha consentito al nostro Paese, in così breve tempo, di constatare i frutti di una politica di accoglienza, di integrazione ma anche di rigore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la questione dell'immigrazione ci pone un problema di contrasto tra buoni principi e cattive leggi: buoni principi che tutti noi, spesso, tendiamo ad avvalorare e sostenere e che l'Europa ci raccomanda

che è stato raccolto nella risoluzione della 3° Commissione, e che ci invita a cooperare con gli altri Paesi dell'Unione europea per un governo europeo dei fenomeni migratori e ad utilizzare appieno gli strumenti della cooperazione allo sviluppo con i Paesi d'origine e di transito.

favorisce, fin dall'inizio, la possibilità che l'immigrato sia di fatto identificato come clandestino e punito come tale e, quindi, altera in modo artificioso un quadro che alcune delle mozioni presentate hanno descritto con notevole chiarezza. Mi riferisco soprattutto alla mozione dei colleghi del Partito Democratico illustrata dal senatore Livi Bacci che, come tutti sapete, è anche un grande esperto di questo argomento. Nella sua prima parte tale

a valutare non solo l'elemento di necessità - la brutale necessità economica che chiede forze di lavoro che la società italiana non produce più ma anche l'elemento di accoglienza e colloquio con energie nuove: la dimensione culturale che ho trovato in quel documento, e che mi è sembrata molto saggia e ben espressa. Di fronte a questa congiunzione tra la necessità e la volontà, alcuni colleghi, in Aula ed anche negli organi di stampa, continuano a riproporre un modello interpretativo basato sostanzialmente sul principio che chi viene da fuori deve interiorizzare i principi della nostra identità. Trovo che la forzatura del ragionamento sull'identità sia qualcosa di ambiguo e che, alla fine, porti a distorsioni di natura politica pericolose. Noi ci rappresentiamo di fronte agli immigrati come un'identità pura. Chissà perché pensiamo al Rinascimento, alle città medievali, ai centri storici ottocenteschi, alla Divina Commedia, anche anche all'ultimo Premio Strega. Ma l'Italia non è solo questo. Cosa offre all'immigrato che viene da fuori e che viene spinto da una necessità impellente e non cancellabile? Guardate che spesso gli offre un quadro dove la maestà della legge è nascosta sotto al tappeto, dove l'effettivo rigore nell'applicazione dei principi costituzionali è dimenticato e vanificato;

solo quello che un politico di qualche anno fa chiamava l'infinita potenza dello Stato. E' invece il contrasto o, peggio ancora, l'inquinamento dell'infinita potenza dello Stato con una capacità della malavita organizzata di tessere reti imprendibili sul territorio. gli immigrati sono doppiamente vittime, perché arrivano spinti da necessità irrimediabili, giungono in una condizione dove la legge dice loro che sono fuori legge, in quella condizione di fuorilegge ricadono sotto il capestro di poteri illegali, che però sono strettamente avvinghiati alla legalità e che con loro capacità pervasiva ed incisiva li sottomettono in un quadro di abiezione che sconfina nella schiavitù. Non possiamo dimenticare, quando noi pensiamo alla nostra identità e ai nostri valori - i nostri famosissimi valori - che in realtà offriamo a questi forzati dell'occupazione necessaria le beatitudini del lavoro nero, che siamo noi a organizzare, che è la società italiana a determinare e ad articolare; non possiamo dimenticare che forniamo loro anche pessimi esempi, che

Vedono che qualche volta i valori della nostra società sono il falso in bilancio, la corruzione in atti giudiziari, il rifiuto della legalità da parte dei potenti e il cammino aperto per quelli che dovrebbero far rispettare la legge e invece, insieme a chi la mina, esercitano un controllo stringente sull'insieme del mercato del lavoro.

sul collo del lavoratore, a cui è stato detto: tu sei un fuorilegge, e allora lavori come fuorilegge e vieni pagato, come fuorilegge, molto, molto meno di tutti gli altri, però dovrai pagare molto, molto di più per l'affitto, perché ti teniamo per il collo.

eccessivamente ottimistico - mi tengo basso - del trattare l'immigrazione come una sorta di adozione a distanza: gli immigrati li adottiamo là dove sono, portiamo loro lo sviluppo, li facciamo lavorare là. Ma se non siamo capaci di portare lo sviluppo a casa nostra, cosa raccontiamo che siamo in grado di determinare meccanismi di sviluppo economico e sociale addirittura fuori dai territori dove esiste la nostra potestà di incidenza? Penso che dovremmo prendere molto più sul serio gli inviti della Comunità europea a trattare la questione con saggezza e umanità, e ritrovo tali princìpi - lo ripeto perché ci tengo - nella relazione del senatore Pisanu. A quel tipo di princìpi dobbiamo attaccarci, ma non dobbiamo produrre leggi proibitive e patogenetiche che costringono vieppiù chi è già vittima ad esercitare un ruolo di vittima doppia o tripla. Ci sono dei fatti che ci dovrebbero far piacere. Il collega della Lega ha sottovalutato il fenomeno della manifestazione di ieri dei migranti. È vero, non erano moltissimi con i nostri metri di giudizio, ed è anche molto probabile che questo sciopero, in quanto artifizio sindacale, sia fallito,

c'era la voce di una giovane esile che parlava con grande efficacia e di cui ricordo soltanto un punto d'applicazione. Si rivolgeva agli ascoltatori mentre il corteo passava per la strada e diceva: signori, ascoltateci, noi siamo umani come voi! Lo diceva con un tono così convincente perché era una voce debole che risuonava fortissima. Queste persone sono la ricchezza del nostro futuro: fanno figli mentre noi abbiamo smesso di farli; lavorano per pochissimo, vivono male eppure si sentono umani; parlano la nostra lingua e qualche volta la parlano anche tra di loro. Credo che nei confronti che nei confronti di questo fenomeno dovremmo rinunciare alla grettezza, all'avarizia, all'insensibilità e riuscire ad esprimere quello che qualche volta, per sbaglio, ci viene meglio del nostro modo di essere. Sforziamoci, però.

una delucidazione. Poco fa, le agenzie hanno dato notizia che lei, signor Presidente, prendendo la parola come Presidente del Senato sull'esclusione delle liste del PdL dalle elezioni regionali del Lazio, ha dichiarato di augurarsi

Presidente, mi permetta di concludere. è un dibattito che non c'entra con questo argomento. Ho fatto l'avvocato per trent'anni e conosco la normativa. Ho parlato di rispetto delle regole. Mi auguro, e lo confermo,

ho detto: «nel rispetto delle regole» e ho detto anche: «La sostanza prevalga sulla forma quando questa non è essenziale». Vi sono casi di essenzialità della forma e casi in cui la forma può essere superata con integrazioni; questo saranno i magistrati ad acclararlo. Do lettura del calendario,

il Presidente del Senato deve tutelare la forma,

La seduta pomeridiana di oggi, per la quale non è previsto l'orario di chiusura, è riservata alla discussione congiunta - fino alle votazioni finali - della risoluzione della Commissione esteri e delle connesse mozioni in materia di immigrazione. Domani mattina la seduta antimeridiana si aprirà con la discussione delle dimissioni presentate dal senatore Nicola Di Girolamo. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo alle ore 12. Per gli interventi che precederanno il voto la Presidenza ripartirà i tempi tra i Gruppi. Qualora non dovessero essere accolte le dimissioni predette, si passerà all'esame delle mozioni concernenti la relazione della Giunta sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero e, in caso di approvazione delle mozioni medesime, 1'ordine del giorno dell'Assemblea si intenderà immediatamente integrato con il seguito dell'esame della citata relazione. Il calendario della settimana corrente prevede inoltre la discussione del disegno di legge collegato in materia di lavoro pubblico e privato, del disegno di legge sul "*Made in Italy*" e di ratifiche di accordi internazionali. Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo, alle ore 16, il Sottosegretario alla Protezione civile renderà un'informativa al Senato sul dissesto idrogeologico, nonché sull'inquinamento del fiume Lambro e del bacino del Po. Successivamente, i rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per 5 minuti ciascuno. Il dibattito sarà trasmesso in diretta televisiva per la durata di un'ora. Resta confermato il calendario della prossima settimana che prevede l'esame dei disegni di legge in materia di legittimo impedimento e di riforma dei COMITES. Nella settimana successiva alla prossima, dal 16 al 18 marzo, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, saranno discussi i decreti-legge concernenti enti locali e competenza delle Corti d'assise, nonché il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza stradale e la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito. Sarà inoltre incardinato, con lo svolgimento della relazione, il disegno dì legge di riforma della professione forense. La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito che 1'Assemblea non terrà seduta nella settimana precedente le elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo. In attesa della definizione del calendario dei lavori delle settimane successive, è stato fin d'ora deciso che nella seduta pomeridiana di martedì 30 marzo inizierà la discussione del decreto-legge sui beni sequestrati alla criminalità organizzata, presentato alla Camera dei deputati.

il nostro voto sul calendario è stato un voto contrario, e lo è stato per una ragione specifica, che è quella che riguarda l'ordine dei nostri lavori della giornata di domani e per l'inserimento al primo punto dell'ordine del giorno, piuttosto che delle mozioni che riguardano la decadenza del senatore Di Girolamo, delle dimissioni presentate dal senatore Di Girolamo successivamente

Quali sono le ragioni per le quali riteniamo che il Senato debba prioritariamente esaminare la decadenza del senatore Di Girolamo? Le riassumerò, ma i colleghi che hanno vissuto questa lunga vicenda - perché di una lunga vicenda si tratta - possono benissimo comprendere comprendere la forza delle argomentazioni. Innanzitutto, c'è un principio di ordine generale, in base al quale vengono discussi per primi i documenti che per primi sono stati presentati. In questo caso, credo che la proposta di decadenza decadenza non possa essere collocata nel momento della presentazione della mozione Sanna, che pure, come abbiamo visto, ha preceduto la mozione Malan e le dimissioni presentate dal senatore Di Girolamo, bensì dobbiamo fare riferimento a quella proposta di decadenza del senatore Di Girolamo che fu avanzata quasi all'unanimità dalla Giunta il 28 ottobre 2008 e il cui *iter*, in maniera assolutamente non solo imprevedibile rispetto alla storia, alla prassi e alle regole che governano questa materia nell'agire della Giunta e nell'agire dell'Aula che furono in quel caso travolte, ma anche - devo dire - con un atto teso a precostituire un precedente pericolosissimo, fu sospeso fino all'esito definitivo e quindi alla sentenza definitiva, al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe deciso sulla ricorrenza del reato che era stato attribuito al senatore Di Girolamo. Una questione delicatissima, che pone innanzitutto una questione di violazione dell'articolo 66 della Costituzione: le Camere hanno competenza, con attribuzione esclusiva, in ordine alla valutazione dei titoli di ammissione ed eventualmente dei titoli di di ineleggibilità che riguardano i propri componenti. L'accertamento della Giunta non è un accertamento che riguardi il ricorrere di una fattispecie piuttosto che di un'altra e un giudizio di colpevolezza su un soggetto piuttosto che un altro: è un accertamento meramente tecnico che viene puntualmente esercitato dalla Giunta anche per il tramite del Comitato inquirente sulla base di tutta la documentazione di cui per scrupolo la Giunta si sia voluta servire servire e che serve esclusivamente a valutare, nell'esercizio di una esclusiva attribuzione, l'esistenza dei titoli per l'ammissione di quel soggetto ad una delle Camere. Con quell'ordine del giorno, abbiamo travolto questo principio dell'articolo 66, costituendo il precedente per cui in tutti i casi in cui ci sia un procedimento penale che riguardi, lambisca, circondi, sfiori la questione che riguarda l'ammissione di un soggetto alla partecipazione alle Camere, il giudizio deve essere sospeso e questo mentre il Regolamento per la verifica, all'articolo 5, prevede che la Giunta possa, esattamente nell'esercizio di quello scrupolo e soprattutto di quella esclusiva competenza, decidere liberamente di sospendere temporaneamente il proprio giudizio per acquisire elementi che possono derivare da un procedimento penale. Esame che, né con la deliberazione del 28 ottobre, né con quella che oggi ci troviamo ad esaminare, la Giunta ha ritenuto di dover mai fare. Il presidente Schifani ha obiettato che ci sono precedenti in materia e ha citato precedenti della Camera dei deputati e un precedente del Senato, che però è contraddetto da un altro precedente. Perché faccio riferimento a questo?

che riguardano la natura squisitamente politica del giudizio operato dalla Giunta e dall'Aula. Ripeto: natura squisitamente politica. politica. La natura squisitamente politica dell'atto ovviamente non prescinde dal contesto istituzionale e politico nel quale le decisioni maturano - se la vogliamo dire tutta - da un deliberato quasi unanime della Giunta, da un atto abnorme, da un'ulteriore pronuncia della Giunta che verrebbe ulteriormente travolta dalla presentazione delle dimissioni del senatore Di Girolamo. Potrei continuare, ma c'è una questione che viene prima di tutto e che riguarda non la mia parte politica, ma - lasciatemi dire - ciascuno di noi e il Senato della Repubblica. È la questione che nel Paese occupa l'attenzione e la preoccupazione di milioni di italiani. Questa vicenda è finita su tutti i giornali d'Italia e potrei dire - ahimè! - del mondo. È una questione che ha seminato sconcerto, preoccupazione, talora ulteriore ripulsa nei confronti delle istituzioni democratiche. E in tutto questo il Senato ritiene di di non dover sanzionare dal punto di vista politico e istituzionale un comportamento che è lesivo dell'onore, del prestigio e dell'autorevolezza del Senato della Repubblica! Dobbiamo anche qui sopire, troncare e ammettere che si discutono solo le dimissioni del collega Di Girolamo per poi, magari, fare domani una bellissima dichiarazione in cui si elogia il senso delle istituzioni e il coraggio civile del senatore Di Girolamo. Colleghi, francamente stiamo maneggiando un bene non disponibile, che non appartiene né alla mia parte politica, né alla vostra. Fatti gravissimi - ripeto: si stanno verificando. Il giudizio non lo facciamo sull'oggi; lo abbiamo già fatto il 28 ottobre del 2008 e lo dico per tutti coloro i quali volessero ravvisare un intento persecutorio nel mio intervento di oggi. Oggi è il momento della responsabilità e della dignità: non è il momento di lasciar correre, di lasciar passare, di mettere la sordina, di far finta che niente sia accaduto.

ancora di dichiarazioni rese da colleghi ovviamente preoccupati per le vicende delle liste, di colleghi della maggioranza che dicono che è inammissibile che le liste le faccia la magistratura. Ma, colleghi, rendetevi conto che con l'ordine del giorno del

cinico e inaccettabile delle regole, delle forme e della stessa dignità delle istituzioni. È per questo, signor Presidente, che io le ho manifestato le ho manifestato oggi la nostra ferma opposizione su questo punto, ed è questa la ragione per la quale voteremo contro il calendario dei lavori da lei proposto.

certamente, per le ragioni illustrate poco fa dalla senatrice Finocchiaro, che per motivi di brevità non intendo ripetere, ma anche per altre considerazioni. La prima fra tutte è la seguente: se un anno fa l'Aula avesse accolto la proposta votata quasi all'unanimità (quindi con il voto dei colleghi in Giunta delle elezioni di maggioranza e di opposizione) e di opposizione) con cui la Giunta ha chiesto la decadenza del senatore Di Girolamo, oggi non saremmo qui ad occuparci di questo problema con argomentazioni che possono apparire cavillose o formali, ma che in realtà sono di natura sostanziale. Verosimilmente, signor Presidente, avremmo potuto inserire nel calendario - come noi abbiamo chiesto - ad esempio, una discussione sui dati dati sulla crisi economica e sull'andamento dei conti pubblici in questo Paese che l'ISTAT, quindi un istituto al di sopra di ogni sospetto, ha fornito, e che sono dati inquietanti in ordine alla disoccupazione, all'aumento della pressione fiscale e al cattivo andamento dei conti pubblici; ad esempio, ci saremmo potuti occupare della relazione, altrettanto seria e altrettanto grave, resa al Parlamento dal COPASIR sulla situazione della sicurezza nel nostro Paese con particolare riferimento al terrorismo internazionale e al terrorismo interno. Invece siamo costretti da una miope ed arrogante decisione della maggioranza di un anno fa, che ha inteso insabbiare questa vicenda, a ritrovarcela qui esplosa, anche da un punto di vista penale, in maniera estremamente seria e grave, e tale da compromettere la credibilità e la serietà delle istituzioni democratiche. Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che il senatore Di Girolamo ha avuto una buona idea nel dimettersi. Certamente questa idea sarebbe stata apprezzata ancor di più se fosse stata in qualche modo frutto esclusivo di una sua spontanea e libera decisione e non della circostanza che

facultato dall'iniziativa che il Presidente del Senato ha assunto, con una lettera indirizzata al Presidente della Giunta delle elezioni, in ordine al riesame della decadenza del senatore Di Girolamo; cioè avremmo apprezzato di più che questa lettera di dimissioni fosse stata presentata non dico qualche mese fa o qualche trimestre fa, ma anche qualche settimana fa. Il punto però è diverso, signor Presidente, ed è il seguente (non voglio ripetere cose già dette): resta una questione molto grave che rischia, se non affrontata in maniera chiara, di precludere alla Giunta delle elezioni l'esame integrale, a norma dell'articolo 66 della Costituzione, delle cause di di ineleggibilità o di incompatibilità con riferimento ai fatti che possono formare oggetto di un procedimento penale.

dei requisiti di eleggibilità di un senatore, se su questi requisiti vi è un'indagine della magistratura e quindi pende un procedimento penale, fino a quando questo procedimento penale non si conclude con sentenza passata in giudicato, su questo tema la Giunta non può decidere. Ora, rimosso il caso Di Girolamo con l'eventuale accoglimento domani da parte dell'Aula delle sue dimissioni, resta in piedi questo indirizzo

a dover discutere di qualche altro caso - ad esempio - di un collega senatore eletto in qualche luogo della Circoscrizione estero, in riferimento ai requisiti - faccio ovviamente ipotesi di scuola, signor Presidente, perché è notorio che i giornali non ne hanno parlato né oggi né nei giorni scorsi e quindi a queste eventuali ipotesi o ad altre, la Giunta per le elezioni non avrebbe alcuna possibilità di svolgere la sua funzione perché vincolata da quel famosissimo ordine del giorno. Che quel famosissimo ordine del giorno sia un problema lo testimonia anche la circostanza che lei, signor Presidente, qualche giorno fa

del senatore Di Girolamo sulla scorta delle nuove risultanze delle indagini penali a carico di detto senatore e di altre settanta persone. Lo testimonia la circostanza che la Giunta, in quel caso, le ha dovuto, suo malgrado, dire di non essere nelle condizioni di poter svolgere alcun esame

identici o analoghi a quello di cui ci stiamo occupando non ha alcuna possibilità di intervenire e quindi - per dirla in modo esemplificativo - ha le mani legate. Ora, proprio per questa ragione, abbiamo depositato una mozione che limita il voto dell'Aula alla revoca dell'ordine del giorno De Gregorio, il quale poteva avere una sua logica - personalmente non l'ho condivisa e non la condivido tuttora - con riferimento a quella circostanza specifica, ma oggi vincola l'attività della Giunta in tutti i casi riguardanti la stessa materia.

trovare il modo di rimuovere quell'ordine del giorno, che non è più di attualità e costituisce un precedente nefasto per l'attività della Giunta di questa e delle prossime legislature, credo possa essere un modo, diverso da quello che magari l'opposizione preferisce, di affrontare la questione e di risolverla definitivamente, lasciando ciascuno di noi ovviamente con con l'opinione che ritiene più opportuna, salvaguardando però l'unità, l'autorevolezza, la credibilità e la trasparenza delle istituzioni, circostanza alla quale ritengo siamo tutti indistintamente legati.

sulla vicenda al voto dell'Assemblea sulle dimissioni presentate dal senatore Di Girolamo.

il dovere ed il diritto di giudicare dei titoli di ammissione di un proprio componente. rispetto al principio costituzionale che assegna alle Camere questa prerogativa alta si è posto quell'ordine del giorno, che chiamiamo De Gregorio dal nome del senatore primo firmatario, che invece applicava, pur non essendo stata invocata da nessuna parte, neanche dal senatore Di Girolamo, la pregiudiziale penale.

degli accertamenti penali vestiti di autorità di cosa giudicata. ha dimostrato molto saggiamente di non condividere questa impostazione contenuta nell'ordine del giorno

di verificare i requisiti di ammissione a questo consesso del senatore Di Girolamo alla luce della nuova documentazione pervenuta. Lei stesso nella lettera che ha inviato, signor Presidente, diceva: «So bene che l'ordine del giorno àncora la decisione all'esito di un giudicato, però essendo pervenuta nuova documentazione, vi invito sollecitamente ad esaminare la questione», ovviamente ben sapendo lei, signor Presidente, che la documentazione pervenuta non era e non poteva essere assistita dall'autorità di cosa giudicata, essendo la richiesta di applicazione di una misura custodiale. Nonostante, però, non si trattasse di questioni e di atti coperti dal giudicato, lei ci ha detto ugualmente di esaminarli perché potevano avere una refluenza e un'importanza sull'eventuale decadenza del senatore Di Girolamo. Quindi, ho interpretato nella sua sollecitazione alla Giunta una correzione rispetto al contenuto giuridico dell'ordine del giorno De Gregorio: ossia la Giunta è investita delle sue prerogative a prescindere dagli atti di cui è in possesso e che deve valutare se siano essi assistiti dall'autorità di cosa giudicata o meno. Questa sua apertura critica, nei confronti di un ordine del giorno che, invece, andava ad impattare con l'articolo 66 della nostra Costituzione oggi viene messa in discussione dall'organizzazione dei nostri lavori. Se lei stesso ci ha detto di valutare le carte anche se non assistite da giudicato, perché tenere fermo un precedente che poi ci ritroveremmo in futuro? Rimuoviamo, dunque, quell'ordine del giorno che lei, signor Presidente, ha dimostrato di non condividere. Rimuoviamo quell'ordine del giorno che vincola l'esercizio delle prerogative al giudicato di un'altra autorità, ossia quella giudiziaria, di modo che non esista un precedente per cui si possa dire che comunque, quando i fatti siano sottoposti alla valutazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 66 della nostra Costituzione, ma siano, al contempo, materia di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria penale,

spazio per la rimozione di quell'ordine del giorno, che oggi probabilmente non è più condiviso, di modo che si elimini un precedente gravissimo che andrebbe in contrasto con la nostra Carta costituzionale e ridia le piene prerogative e sovranità e dignità delle immunità parlamentari, così come disciplinato dal nostro Regolamento e nel rispetto della Carta costituzionale. Rimuova quel precedente infausto. Ha dimostrato di volerlo fare; dia corso a questa rimozione nell'interesse della nostra Assemblea; eviti cioè un nefasto precedente.

sicuramente strumentali e anche fuori luogo. Capisco che siamo in campagna elettorale, però è anche vero che il tema dev'essere affrontato per quello che è.

del senatore Di Girolamo, eletto nelle liste del Popolo della Libertà. Loro invece chiedono il voto per la decadenza.

senatore della Repubblica sia se votiamo per le dimissioni sia se votiamo per la decadenza. Da domani pomeriggio il senatore Di Girolamo dovrà rispondere dovrà rispondere di quello che ha fatto ai magistrati e molto probabilmente domani sera il senatore Di Girolamo dormirà per la prima volta nella sua vita in carcere perché sarà arrestato. Questi sono i risultati del voto che saremo chiamati domani a dare: sono, quindi, assolutamente identici,

sulle dimissioni le stesse non venissero accolte dall'Aula, visto che è un voto segreto, noi confermiamo il voto per la decadenza del senatore Di Girolamo nella mozione successiva. Dunque, non cambia assolutamente nulla. Dispiace vedere ancora una volta in quest'Aula, visto che siamo in campagna elettorale, chi fa un falso moralismo perché, se vogliamo parlare di fatti di cronaca che riguardano anche i rappresentanti

ebbene, sia il Partito Democratico, sia l'Italia dei Valori, sia l'UDC in molte Regioni di questo Paese candidano inquisiti e hanno candidati Presidenti che sono stati rinviati a giudizio. *(Applausi dal

Le faccio presente che fra le vostre fila avete rappresentanti del territorio che sono stati inquisiti, rinviati a giudizio per falso, abuso d'ufficio, corruzione, concussione, associazione a delinquere.

parliamo di cose concrete. Domani voteremo le dimissioni del senatore Di Gregorio... C'è poco da ridere; potrei fare l'elenco delle persone (ma, come dicevo, non lo farò) che sono presenti in questo Parlamento perché, grazie all'immunità, evidentemente possono...

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiarire in primo luogo che il nostro Gruppo ha presentato una mozione

della giustizia ordinaria era certamente condizionata da una conseguenza ulteriore, che non era solo la decadenza ma l'arresto

Abbiamo maturato il convincimento di presentare una mozione - che è agli atti - per dire che quella richiesta di sospensione va sospesa: oggi in un contesto diverso, con accuse diverse che poi sarà la magistratura a valutare, è plausibile, di fronte a fatti diversi, di grande rilevanza penale, che anche quell'indirizzo non fosse vero. Peraltro, aggiungo - e lo dico senza bisogno di interruzioni - che su indirizzi e vicende di voto all'estero la confusione regna sovrana, al punto che il nostro Gruppo condivide e si fa promotore di iniziative tese non a negare il diritto costituzionalmente sancito di avere nelle Assemblee parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero (lunga e giusta battaglia discussa tante volte in Parlamento), ma di rivedere le modalità di elezione - questa è la verità - che è un'esigenza diffusa.

ho letto giorni fa sull'«Avvenire». Faccio da cronista, non ne traggo conclusioni o giudizi: non è questa la sede, né il momento. Si tratta di colleghi di Camera e Senato, appartenenti a Gruppi della sinistra, e le discussioni vertono sui plichi, i pacchi, i voti e le preferenze, riferiscono di questa casistica. Credo che si debba riflettere al fine di definire procedure elettorali certe, perché poi quando il collegio è l'Oceania o l'America Meridionale, mi rendo conto che non è molto facile. Ma così le cose non vanno bene, per una molteplicità di casi. Abbiamo quindi presentato una mozione relativa alla sospensione di quella decisione che riguarda quella vicenda e che, a nostro avviso, non costituisce alcun precedente, perché fu una decisione che riguardava quella vicenda, condizionata non solo da una richiesta di decadenza, ma da conseguenze che in quel momento apparivano, almeno alla maggioranza dell'Assemblea, eccessive rispetto a quei fatti, non a questi fatti.

Si considerò addirittura autentica quella comunicazione arrivata sul momento e si votò sulle dimissioni dell'onorevole Cesare Previti. C'è ancora un altro precedente,

allora ebbe a conoscere delle dimissioni dell'onorevole Crippa in corso di dibattito e l'allora Presidente della Camera dei deputati, in data 18 dicembre 1993, disse che per un principio di economia procedimentale era corretto

Quindi, riteniamo che la procedura seguita dal Presidente del Senato non solo sia da sostenere, ma non potesse essere diversa, perché si rifà a precedenti di decisioni assunte dal presidente Bertinotti, dal presidente Pera e dall'allora presidente della Camera Giorgio Napolitano. Questo per essere molto chiari. chiarito che la nostra mozione sulla sospensione della sospensiva c'è: poi ne discuteremo, ma per noi quella questione è chiarita e risolta perché era riferita a quel caso e non costituisce un precedente per altri casi.

questo modo. A nostro avviso, proprio rispetto alla materia che discutiamo e alla vicenda in sé, mentre se tornassimo a discutere della decadenza, decideremmo sull'indirizzo, vero o falso, domani - come mi auguro, dato che voterò a favore delle dimissioni Di Girolamo - ritengo che la situazione imponga al Senato, a tutti noi, una valutazione diversa. Il senatore Di Girolamo ha presentato le dimissioni ieri, in relazione a vicende di carattere giudiziario che sono ben più gravi e complesse di quelle che discutevamo in merito all'indirizzo. Quindi, se si vuole sottolineare la gravità di quanto accaduto e dare a questa vicenda

che lo attendono al momento), ritengo che proprio le dimissioni siano collegate a queste vicende, perché arrivano dopo di esse. Pertanto, se vogliamo dare un segnale politico, è proprio il voto favorevole alle dimissioni dopo queste ulteriori accuse che assume un grande valore morale, non il tornare sulla vicenda precedente. Non eludiamo alcun nodo e condividiamo la proposta di calendario. Ho citato alcuni precedenti autorevoli in realtà di fatto che riguardano casi diversi tra loro, ma nei quali Presidenti diversi, appartenenti

Signor Presidente, colleghi, signor ministro Maroni, penso che la relazione fatta all'inizio di questa discussione dal presidente Pisanu offra un'occasione politica importante: l'occasione per un confronto che cerchi di uscire dalla ripetizione di un conflitto tra parti che rifiutano di ascoltarsi per aprire una fase diversa

sostanzialmente una visione di chiusura rispetto ad un processo così importante. Il senatore Pisanu ha detto in Commissione esteri e ha ripetuto qui che l'unica alternativa all'immigrazione irregolare è l'immigrazione regolare: questa è la strada sulla quale è necessario camminare per tante ragioni. Sappiamo che le politiche di chiusura che sono state adottate fino ad oggi hanno, certo, ottenuto dei risultati. Naturalmente il ministro Maroni può dire che gli sbarchi e le partenze dalla Libia sono cessate, e questo è sostanzialmente vero. Ma le chiedo, signor ministro Maroni: degli 80.000 visti 80.000 visti dati in Ucraina per l'ingresso in Italia nel 2008, quanti si sono trasformati in una permanenza che è andata al di là dei limiti del visto? E dei circa 400.000 visti che sono stati dati in Russia, quanti rimangono oggi come *overstayer*? Siamo di fronte ad un problema che ha queste dimensioni, che ha queste caratteristiche.

e che addirittura l'11,3 per cento degli occupati è costituito da immigrati: ciò a segnalare che anche durante il periodo di crisi, nonostante le grandi difficoltà che attraversa il mondo dell'occupazione, il fenomeno dell'immigrazione continua e si accentua. se il problema è quello di come costruire immigrazione regolare governando i flussi, i flussi, vorrei richiamare tre questioni che già il collega Livi Bacci ha affrontato nella sua relazione e sulle quali chiedo se è possibile un confronto di tipo diverso. Prima questione. senatore Livi Bacci ha detto: noi pensiamo che sia necessario, se vogliamo promuovere l'immigrazione regolare ed affrontare questo grande problema, promuovere permessi di soggiorno per ricerca di lavoro,

definendo regole e criteri precisi, permetta di affrontare tale strada? È possibile farlo, ad esempio, prevedendo all'inizio che una simile possibilità riguardi una quota limitata di persone, seguendole con attenzione e sperimentando che ciò avvenga promuovendo regolarità e non irregolarità?

contribuisce a costruire ordine e a costituire elementi di stabilità e contribuisce a un inserimento più funzionale, più organico, migliore delle persone nella nostra società?

il problema del diritto all'asilo e alla protezione umanitaria di coloro che possono, perché il diritto internazionale glielo garantisce, avanzare tale richiesta. come è possibile garantire che una persona che ha diritto di avanzare la richiesta di asilo e di protezione umanitaria possa farlo senza mettere a rischio la propria vita, senza mettersi nelle mani dei mercanti e di coloro che praticano la tratta di essere umani? È possibile o no su questo punto sperimentare strade

e la ricerca di soluzioni per garantire in modo regolare e legittimo l'esercizio del diritto alla protezione umanitaria)

il senatore Pisanu. Penso che, se ci fosse il coraggio di partire dalla relazione del senatore Pisanu per proporsi di cambiare i rapporti tra di noi e di compiere

di non ripetere semplicemente le sue convinzioni, ma di misurarsi su un terreno nuovo come quello proposto nell'intervento che introdotto la nostra discussione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di non tediare i colleghi rimasti in Aula ripetendo ciò che ho già detto nell'illustrazione della mozione presentata dal mio Gruppo. Cerco di prendere una strada diversa e forse anche più breve. Una parola soltanto sull'osservazione, molto cara ad alcuni colleghi, circa la rilevanza della popolazione carceraria immigrata, che sarebbe la dimostrazione di una sorta di tendenza irresistibile alla devianza sociale da parte degli immigrati. Ci sono tanti carcerati immigrati: questo - essi sostengono - prova, al di là di ogni dubbio, che siamo di fronte a dei delinquenti nati. Si potrebbero eccepire molti elementi in contrario, ne cito solo uno: la tradizione giuridica che in Italia ha portato letteralmente a demolire il processo penale, come molti giuristi e molti magistrati possono testimoniare con cataste di pubblicazioni. Questa demolizione del processo penale ha avuto un risultato del tutto asimmetrico: proteggere gli imputati di rilievo, i potenti, i colletti bianchi, rendendo irraggiungibili e inattingibili dalla giustizia coloro che delinquono in modo elegante, con moltissimi soldi e moltissimo potere. È ovvio che questa sorta di sottrazione preventiva alla severità della legge di tutti costoro determina una sperequazione: alla fine, in galera ci vanno solo i poveracci, che non hanno soldi, che non possono pagarsi gli avvocati bravi e che è facile prendere. Ovviamente lo spacciatore di quartiere è facilissimo da prendere, mentre sembra che in Italia

Penso che in Italia, e anche a Roma, siano già in atto straordinarie

le persone si integrano nella nostra vita, siamo tutti buoni e ci vogliamo bene. La società - grazie al cielo - è conflitto, è esercizio della capacità del conflitto reciproco: una società che non abbia conflitto è una società morta.

un'esperienza che è cominciata, come sempre succede in questi casi, da piccoli *incipit*, da tentativi artigianali e che alla fine ha prodotto un fenomeno di natura musicale straordinariamente brillante,

strumenti del tutto inusuali (non parlo di orchestre che eseguono la Nona di Beethoven: ci sono strumenti originali delle varie culture e dei vari paesaggi geografici e culturali del mondo), e che si è realizzata

talvolta fanno quasi finta di litigare nella realizzazione dei loro a solo nell'insieme orchestrale, con una sorta di dialettica che è anche spiritosa e ironica. desidero concentrare l'attenzione soprattutto sulla potenza della scuola intesa in senso costruttivo. Molti immigrati fanno, come ci ricorda il senatore Livi Bacci, molti più figli degli italiani e molti di questi figli vanno a scuola, ma non tutti. Penso che, molto più delle misure repressive, di gran lunga la più possente arma

Questo è l'elemento fondamentale: lo studio è l'applicazione, ma l'accesso alla conoscenza è quello a cui tutti davvero hanno diritto, perché non sapere è la cosa peggiore che possa capitare a qualsiasi cittadino: è una cosa che rende minoritari, insufficienti ed anche inutili. Sapere, naturalmente, è sapere di non sapere, è sapere che bisogna continuamente avere un atteggiamento di ricerca, di approfondimento, di critica. Quindi, il diritto alla conoscenza è la cosa fondamentale. Noi ci dovremmo impegnare su questo fronte, e dovremmo farlo con un senso quasi di allegria sociale, perché leggo, ad esempio, sui giornali che l'atteggiamento di questa maggioranza nei confronti di tale fenomeno riesce a partorire soltanto la terribile definizione del limite degli studenti di provenienza esterna come quota che non può essere superata. Vedete con che mentalità malata ragioniamo su questo argomento?

Quando mai avremo davvero la dimostrazione che sono quelle percentuali di immigrati che minano la forza e la capacità di "super organismo" che spesso hanno le classi quando sono ben riuscite? Questa idea della solidarietà reciproca, ma anche l'idea della critica, l'idea dello sfottimento del compagno, l'idea della presa in giro: tutto fa società.

negli ultimi vent'anni ha insegnato storia dell'arte, una materia bellissima che riesce ad apparire fascinosa, se la si sa insegnare, a tutti e non solo agli studenti italiani.

sissignore! E quando i ragazzi di quella stessa classe non avevano capito bene qualcosa di Piero della Francesca o di Masaccio, la studentessa cinese era capace di spiegare meglio ai suoi compagni di classe per far loro capire quello che non avevano capito. Possono essere migliori di noi: questo è il punto. Anzi, dobbiamo augurarci che possano essere migliori di noi. Sono un regalo per la nostra società. Arrivano, sono freschi e hanno voglia di imparare. Perché dobbiamo avere questo atteggiamento di proibizione? Facciamoli crescere, facciamoli studiare. Miglioreranno anche noi.

giungiamo oggi per la prima volta - e per questo ringrazio sinceramente il senatore Pisanu e il senatore Livi Bacci - a una discussione generale sull'immigrazione, come è giusto che sia. Infatti, è proprio l'accettazione del fenomeno migratorio come bisogno reciproco delle nostre società e di chi compie questa scelta (e quindi il riconoscimento come fenomeno strutturale) alla base di un'impostazione comune, mettendoci così finalmente al passo con gli approfondimenti e l'azione delle istanze europee. Integrazione, principio di legalità e di non discriminazione, ordine pubblico e diritti di cittadinanza sono i principali argomenti di discussione che stanno affrontando la politica europea e quella internazionale e che naturalmente deve affrontare anche il nostro Paese. La scelta dell'Unione europea, con i suoi primi atti in materia di politica comune dell'immigrazione, è concepita sulla sostanziale differenza fra immigrazione subita e scelta; una differenza, quindi, e non una contrapposizione che preluda ad interventi di maggior efficacia e coerenza. Un approccio che aiuta a sviluppare un metodo di lavoro integrato che investe problematiche di politica estera, cooperazione, politiche ambientali, commercio internazionale, sicurezza, giustizia, libertà e cittadinanza e che deve concorrere alla definizione di modelli nazionali condivisi. Inoltre, affrontare il problema dell'immigrazione in modo solidale significa che qualsiasi approccio globale non può ignorare i fattori di spinta che inducono le persone a intraprendere, anche con modalità tragiche, la strada dell'esodo forzato. Per questo c'è bisogno di ridare respiro e dignità ai piani di sviluppo e di investimento nei Paesi di origine e di transito, anche facilitando, come si è detto, le rimesse dei migranti verso i loro Paesi di origine. C'è bisogno di ridare respiro e dignità alle politiche sui rimpatri, così come previsto dalla direttiva omonima che questo Governo continua a non voler recepire nella sua totalità. C'è bisogno anche di politiche commerciali e agricole che promuovano le opportunità economiche e di lavoro *in loco*, nonché di politiche che sviluppino lo stato di diritto e affermino nella pratica l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Contestualmente voglio sottolineare che l'Europa, nel mentre non contempla la regolarizzazione di massa degli immigrati illegali e irregolari, non considerandola una risposta adeguata, allo stesso tempo favorisce la regolarizzazione mirata, come previsto nella direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che prevede anche la regolarizzazione per coloro che contribuiscono all'emersione di fattispecie criminose legate all'immigrazione. quella stessa direttiva respinta in quest'Aula appena 15 giorni fa da questa maggioranza di Governo. Cari colleghi, per governare l'immigrazione "di qualità" - e per qualità intendiamo l'immigrazione legale c'è bisogno di rafforzare gli accordi di bacino e gli accordi bilaterali tra i Paesi di immigrazione e quelli di emigrazione, di scegliere come strategie di sviluppo interventi di sostegno alle emergenze e ai profughi e di collaborare con i Paesi di transito. In sostanza, è necessario, come ricordavano altri colleghi, che il nostro Paese persegua coerentemente, attivamente e responsabilmente, investendo risorse materiali e umane, l'obiettivo di un governo europeo dell'emigrazione. Si tratta perciò di consolidare una politica di immigrazione che instauri un giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona. Caro ministro Maroni, colleghi della maggioranza, se non procediamo celermente su questa strada corriamo il rischio di un'ulteriore emarginazione del nostro Paese, già sotto osservazione per l'approvazione delle norme contestate in materia di sicurezza e per i noti fatti di Rosarno.Infatti, la richiesta italiana di una politica comune sull'immigrazione appare in Europa sempre di più strumentale ed ambigua, quando non pretestuosa, e rischia di relegarci in un'area di continuo sospetto sul nostro europeismo. Partendo allora dalla nostra esperienza nazionale, non credo di esagerare nell'affermare che in questa travagliata fase interna ed internazionale emerge un bisogno di più Europa. Fatti come l'euro, l'allargamento, il Trattato di Lisbona hanno creato per la prima volta nella storia dell'integrazione europea questo bisogno che si sta manifestando nel momento più difficile, quello di una crisi profonda che non è tanto quella dell'Europa e delle sue istituzioni, ma quella dello Stato nazionale, arrivato all'ultima fase di un declino che si trascina da decenni e che denuncia l'assoluta incapacità a fronteggiare le sfide del presente e quelle molto più impegnative del futuro.

che si trova a confrontarsi con il tema della coesistenza tra valori, princìpi e culture diverse su cui la classica nozione di Stato-Nazione si è strutturata. Un cammino, questo, necessario per alimentare su basi nuove la solidarietà e la responsabilità non solo all'interno dell'Unione, ma anche nella sua proiezione esterna. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole del presidente Pisanu nel momento in cui ci ha relazionato sulla risoluzione approvata dalla Commissione affari esteri. Al di là Al di là dell'enfasi e al di là dei numerosi punti di convergenza che ritroviamo nelle diverse risoluzioni, parecchi dubbi cominciano ad offuscarmi la mente e a farmi credere che forse molta retorica e molte strumentalizzazioni vengono fatte di questo argomento. Sappiamo quanto a lungo il dibattito sull'immigrazione abbia risentito degli imperativi di una demagogia supponente, che pretendeva di ridurre l'intera questione alla favolistica contrapposizione di buoni da una parte e cattivi dall'altra, cioè all'antagonismo tra la cosiddetta apertura al diverso, propria delle coscienze illuminate, e le presunte fobiche chiusure manifestate da retrivi egoisti. I documenti su cui ora siamo chiamati ad esprimerci ci riportano con i piedi per terra, meglio - direi - con i piedi in Europa; questo perché negli altri Paesi del vecchio continente il problema immigrazione viene affrontato con una maturità - è stato ricordato già in quest'Aula - che a casa nostra ha faticato ad affermarsi, pur trovando corrispondenza nella lungimirante concretezza delle proposte espresse dalla Lega Nord. Permettete questa rivendicazione; non amiamo le autocelebrazioni, ma qualcosa va pur riconosciuto a chi ha pagato un prezzo salato in termini di linciaggi mediatici e gratuite accuse di razzismo per aver affermato ciò che in Italia veniva bollato alla stregua di eresia, mentre negli altri Paesi dell'Occidente appariva e appare come buonsenso, realismo, premura per il bene comune, per aver affermato cioè che l'immigrazione va governata e che il fenomeno della clandestinità richiede prevenzione e repressione. Pensiamo, a proposito di certe animose quanto infondate campagne, ai fiumi di inchiostro e di parole profusi in occasione dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina nell'ordinamento italiano. I Soloni del pensiero politicamente corretto e del buonismo pretestuoso si strappavano le vesti, incolpandoci di estraniare il Paese dal consesso delle Nazioni civili. inesattezze macroscopiche, poiché l'immigrazione clandestina è trattata come reato dai Paesi più sviluppati, a cominciare dalle principali Nazioni europee dove viene punita con pene detentive, a differenza della mera sanzione pecuniaria oggi prevista in Italia; e non voglio ricordare i vari casi già citati dei Paesi europei. Ho fatto riferimento alla surreale diatriba innescata dall'introduzione del reato di immigrazione clandestina in Italia, non solo per sottolineare la strumentalità di certi anatemi indirizzati al nostro movimento, ma anche per sgomberare il campo da qualsiasi ambiguità nel momento in cui si trattano temi come questo atto comunitario n. 17 esaminato dalla 3a Commissione. Il titolo recita - badate bene - «Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie». Ebbene, si prenda atto che tale approccio globale, manifestato dalla prassi e dal diritto degli Stati europei, non consente l'impunità dei clandestini e dunque pone precisi limiti all'accesso. In quest'ottica il Gruppo della Lega Nord non può che identificarsi nel giudizio di piena condivisione espresso dalla Commissione, la quale ribadisce istanze che ci appartengono e che trovano conferme nelle scelte europee di chi rifiuta l'anarchia degli ingressi sul proprio territorio, magari corretta dalla pratica ipocrita delle periodiche sanatorie. Sottoscriviamo, dunque, i punti della risoluzione che partono dalla premessa irrinunciabile di organizzare l'immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità dell'accoglimento stabilite da ciascun Stato membro. Dal riconoscimento di questa priorità discende l'espressa determinazione di combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno nel loro Paese d'origine o in un Paese di transito degli stranieri in posizione irregolare, e di rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere. Sottoscriviamo - dicevo - e puntualizziamo, perché la mozione del nostro Gruppo intende porre l'attenzione del Governo in momenti qualificanti di queste opzioni. Si tratta, infatti, di perseverare nella strada già intrapresa con successo sullo scenario internazionale con gli accordi di cooperazione, che ottimi risultati hanno conseguito sul fronte degli sbarchi irregolari - Lampedusa ne è una testimonianza e proseguendo con decisione nelle politiche di più recente adozione, segnatamente l'attuazione del cosiddetto permesso a punti, rivelatosi efficace strumento di integrazione nei Paesi che l'hanno adottato. Ultima, ma non meno importante questione, toccata tanto dalla risoluzione della Commissione che dalla mozione presentata dalla Lega Nord, è l'urgenza di riconsiderare l'apporto di manodopera immigrata nel contesto dell'attuale crisi economica. Da un rapporto pubblicato in questi giorni dalla camera di commercio di Monza e Brianza viene rilevato - cito testualmente - che in Lombardia, con la crisi, non sono stati assorbiti nel mondo del lavoro dalla richiesta delle imprese oltre 14.800 dipendenti immigrati, la metà dei quali riguarda Milano. Analoga tendenza viene evidenziata anche in altre Regioni. Nelle attuali condizioni di saturazione del mercato mantenere gli stessi flussi migratori significa consegnare migliaia di persone alla disoccupazione o al più bieco sfruttamento. Non vorremmo insomma che, in nome di un malinteso buonismo, si calpestassero le aspettative degli stessi stranieri e i valori di una società progredita, che dovrebbe farsi garante di quelle giuste condizioni di lavoro proclamate come irrinunciabili sin dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

troppe volte in questi anni il nostro Paese ha affrontato il problema dell'immigrazione con un approccio di emergenza. Quasi sempre il legislatore ha fatto leggi, il Governo ha operato ed il sistema Paese ha affrontato uno dei grandi problemi della società contemporanea sotto la spinta di emozioni forti. Troppo spesso queste emozioni, frutto anche di preoccupazioni, di paure, di ansie pienamente comprensibili e spesso giustificate, si sono trasformate in paure irrazionali, in sentimenti incontrollabili, talvolta alimentati ad arte da chi ha intuito e compreso che sulle paure e sulle insicurezze si può creare facilmente un consenso elettorale; assai più facilmente che affrontando, senza formule magiche o promesse "un tanto al chilo" problemi troppo complessi e delicati per essere liquidati con dei facili slogan di cui ho sentito, anche in qualche intervento di questa sera, qualche eco. È mancata nel Paese nel corso degli anni una visione lunga e ampia del problema. È mancata la consapevolezza che la società italiana tra vent'anni, quando i ragazzi che nascono oggi saranno maggiorenni, dipenderà tanto, molto, dalla capacità che avremo oggi, domani, di avere un progetto serio, coraggioso, realistico, ma lungimirante per affrontare il problema dell'immigrazione e della presenza nella società italiana di una parte consistente e crescente di popolazione proveniente da altri Paesi. Come Ministro dell'interno nel 2000 e nel 2001 ho dovuto affrontare anch'io vere e proprie emergenze e so che queste ci sono e ci saranno. E so anche che le emergenze si affrontano e che talvolta occorre determinazione. Ho affrontato il dramma dell'immigrazione incontrollata proveniente dall'Albania dopo una vera e propria dissoluzione di quello Stato. Abbiamo affrontato l'emergenza, contrastato la criminalità che gestiva il *business* del traffico degli esseri umani. Proprio in questi giorni, ministro Maroni, lei ricorderà che ricorrono i 10 anni da quella operazione che si può definire sicuramente una delle più efficace azione di polizia coordinate sul territorio. Mi riferisco alla cosiddetta Operazione primavera, che ha letteralmente estirpato una crescente organizzazione criminale che, nata dal contrabbando di sigarette, stava organizzando traffici di armi, droga, esseri umani, donne, bambini ed immigrati clandestini. Il presidente Napolitano, nel 1997 ministro dell'interno, aveva dovuto affrontare l'emergenza sbarchi proveniente dalla Tunisia. Egli aveva inaugurato la stagione degli accordi di cooperazione bilaterale e degli accordi di riammissione che si sono rivelati, senza dubbio, la strada più efficace nel contrasto all'immigrazione clandestina. E nessuno meglio di noi sa che una seria politica per governare il fenomeno dell'immigrazione ha bisogno anche di un efficace, fermo e razionale contrasto all'immigrazione clandestina, le cui pratiche generano ripeto - le persone che sono costrette a ricorrervi una condizione di drammatica debolezza e di vulnerabilità. avete commesso, colleghi della maggioranza, soprattutto alcuni di voi, l'errore ingiusto e ingiustificabile di considerare e presentare gli immigrati, anzitutto quelli clandestini, come pericolosi criminali. Molti di loro sono quelle donne e quegli uomini a cui abbiamo affidato tutti noi, tra una sanatoria e l'altra, i nostri figli, i nostri anziani, le persone deboli, i nostri lavori più duri nelle campagne e nelle fabbriche, lavori che nessun italiano accettava. La stragrande maggioranza di queste persone ha impegnato tutti i propri beni, costati anni di duro lavoro, per comprare un viaggio infernale e pericoloso per raggiungere il nostro Paese, inseguendo un sogno, il sogno di un lavoro civile e di una vita dignitosa. Altro che criminali! E con i criminali veri, magari, non siamo sempre stati capaci di dare la risposta necessaria, dura e inflessibile. Ora nella risoluzione presentata dalla Commissione esteri con la firma autorevole del collega Beppe Pisanu, che questi problemi ha seguito con la prudenza e con la competenza che tutti gli riconosciamo, emerge una più equilibrata impostazione. Si respira finalmente un'area un po' diversa da quella degli slogan semplicistici e talvolta beceri; si respira la consapevolezza che il problema da affrontare è complesso e richiede azioni complesse, alcune delle quali di lunga durata e molte da porre in essere in un contesto internazionale. I dati demografici che in più occasioni, con l'autorevolezza dello studioso internazionalmente riconosciuto, il collega Livi Bacci ha illustrato, dicono con grande chiarezza che nel Sud dell'Europa la leggerissima crescita della popolazione sarà sostenuta solo dall'immigrazione, che nel nostro continente l'età media della popolazione continuerà a crescere vertiginosamente. In pochi decenni l'Europa è passata dal 20 per cento della popolazione del pianeta all'8 nel contempo, quella africana è passata dall'8 per cento a oltre il 20 per cento nell'arco di poco più di una generazione. Il tasso di natalità, soprattutto nell'Africa sub-sahariana, continuerà a essere altissimo e la pressione demografica, senza politiche di cooperazione da localizzare nei Paesi ad alto tasso di natalità e a bassissimo reddito medio *pro‑capite*, è destinata a diventare incontenibile, spingendo milioni di persone disperate verso un sogno - ahimé! - assai diverso dalla realtà. Di questa esigenza di guardare all'emigrazione con la consapevolezza di far fronte ad un problema complesso e delicato che esiste da sempre e di affrontarlo anche sperimentando soluzioni innovative, coraggiose e pragmatiche vi è traccia nella risoluzione della Commissione. La mozione n. 245 dei colleghi del mio Gruppo, di cui è primo firmatario il senatore Livi Bacci, affronta con intelligenza e lungimiranza il problema e suggerisce linee di tendenza che andranno approfondite, seguite e tradotte in un provvedimento legislativo, in direttive e in azioni della pubblica amministrazione. Colleghi, nei prossimi anni ci attende un serio e duro lavoro che dovrà tener conto sicuramente delle preoccupazioni, della domanda di sicurezza, della valorizzazione dell'identità della nostra gente, ma che nel contempo dovrà essere idoneo a trasformare con coraggio un problema in un'opportunità, a trasformare in energia vitale la voglia di riscatto, a investire in modo qualificato e produttivo risorse nelle politiche scolastiche e formative ed ad affrontare i nodi delle politiche locali necessarie per assicurare equilibrio nelle nostre città. Presidente e signor Ministro, da oggi, come speriamo, diventerà veramente prioritaria questa scelta di fondo, per il nostro Paese si aprirà una soluzione nuova, all'altezza di un Paese che ha fatto sempre della sua posizione geografica un punto di forza e di apertura. La politica dei ponti levatoi alzati, del filo spinato e delle cannonate, infruttuosa a fermare l'immigrazione clandestina con i rulli di tamburo, è - speriamo definitivamente - seppellita. Una pagina di civiltà e insieme di tutela degli interessi essenziali del nostro Paese potrà essere scritta. Noi, signor Presidente e colleghi, vigileremo perché quella di oggi non resti una pagina isolata di buon senso.

ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito esprimendo posizioni, proposte, indicazioni di

con le politiche di rigore che il Governo ha adottato e con interventi importanti e significativi sul piano dell'integrazione di chi viene nel nostro Paese, o in Europa, per lavorare e non per delinquere.

La legge Bossi-Fini si fonda su un principio considerato innovativo quando venne introdotto ed oggi ripreso dalle legislazioni di tanti Paesi europei:

mi pare che la Costituzione italiana, proprio all'articolo 1, parli di Repubblica fondata sul lavoro. Questo principio è talmente valido che è stato recepito dalla legislazione di molti Paesi: da ultimo, qualche mese fa, dalla legislazione che ha modificato la legge sull'immigrazione della Spagna. Il governo Zapatero ha dunque accolto nell'ordinamento spagnolo proprio il principio fondamentale contenuto nella legge Bossi-Fini.

proponendo, per esempio, la concessione di visti per ricerca di lavoro, con garanzie finanziarie o di *sponsor* istituzionali. Ricordo che il cosiddetto *sponsor,* i permessi di soggiorno per ricerca di lavoro vennero introdotti dalla legislazione precedente ed eliminati proprio dalla legge Bossi-Fini, e credo che questo sia stato un vantaggio che ha determinato il ridursi di

termine che viene spesso usato per contestare iniziative legislative della maggioranza, che non so bene cosa voglia dire. Ricordo che il Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, approvato dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo, chiede agli Stati membri di non procedere proprio a regolarizzazioni. Per quanto riguarda la proposta di riformare la normativa sulla concessione della cittadinanza

ho già espresso e confermo il mio parere assolutamente contrario. L'efficacia dell'impianto legislativo è confermata anche dai risultati che sono stati ottenuti nel contrasto all'immigrazione clandestina, grazie alle leggi vigenti

i casi di segnalazione e di denuncia di immigrati clandestini nel nostro territorio. Grazie a queste misure, grazie alla legge Bossi‑Fini e all'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, i risultati sono evidenti: nel 2008 erano sbarcati

fortemente negativa nei confronti dell'immigrazione in generale, cioè il problema degli sbarchi e dei barconi che arrivano in Italia, abbiamo lavorato intensamente, e i risultati sono assolutamente positivi. Il Centro di Lampedusa è praticamente vuoto,

Nel 2008 rispetto al 2007 il calo era stato dell'1 per cento; nel 2009 rispetto al 2008 è stato del 13,9: il doppio del calo complessivo dei reati. Credo che abbia influito molto positivamente sul calo dei reati commessi dagli stranieri

di amicizia, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008. In questo accordo, che ha portato i risultati che ho citato, le parti si impegnano a intensificare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina (articolo 19). Pertanto, i richiami contenuti nelle mozioni affinché si proceda a stipulare con la Libia accordi in questa direzione non sono accoglibili perché questi accordi sono già in essere e nel testo del Trattato di amicizia se ne parla esplicitamente. Lo stesso articolo 19 del Trattato stabilisce l'impegno delle parti a collaborare alla definizione di iniziative, sia bilaterali sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori; ricordo che la Libia è un Paese di transito e non di origine. Queste disposizioni sono da leggersi in connessione con quanto previsto dall'articolo 6 dello stesso Trattato di amicizia sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sancendo l'impegno delle parti ad agire conformemente agli obiettivi ed ai princìpi della Carta ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ricordo che la Libia ha firmato e ratificato la Convenzione dell'Unione Africana del 1969. Questo trattato, non solo è complementare alla Convenzione di Ginevra, ma rispetto ad essa è di gran lunga più esteso, in quanto impegna la Libia a garantire protezione, non solo ai perseguitati, ma anche alle vittime di invasioni, di guerre civili e di altri eventi di ben più ampia portata rispetto, addirittura, a quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra. la Libia ricopre, attualmente, la carica di Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e che ha presieduto, nel 2003, la Commissione delle Nazioni Unite per il rispetto dei diritti umani.

si è trattato di nove operazioni di riaccompagnamento in Libia per complessive 834 persone. A fronte di una riduzione di sbarchi pari a 834 sono quelli che sono stati riaccompagnati in Libia. Questo, però, è avvenuto in un quadro di assoluta legalità nazionale e internazionale. Nel corso delle operazioni di riconsegna dei clandestini nei porti di provenienza, quelli libici appunto, si è sempre agito in conformità con il principio del *non-refoulement*, perché non è stata negata a nessuno dei clandestini intercettati la possibilità di chiedere asilo. Né alcuno degli stranieri intercettati e soccorsi, una volta saliti a bordo delle navi italiane, ha manifestato la volontà di chiedere asilo. I responsabili delle forze intervenute hanno riferito che durante le operazioni di soccorso in alto mare, durate in media 10 ore, gli stranieri intercettati riaccompagnati) non hanno chiesto alcuna forma di protezione internazionale, né hanno fatto sapere di essere perseguitati nel loro Paese. Al contrario, nei pochi casi in cui gli stranieri hanno chiesto la protezione internazionale, la riconsegna alla Libia non è stata effettuata e gli immigrati sono stati accompagnati sul territorio nazionale per avviare le procedure previste. Le operazioni di riconsegna alla Libia sono avvenute in una cornice di legalità internazionale, anche perché, in applicazione del principio di cooperazione tra Stati internazionalmente riconosciuto, l'unità navale di uno Stato può fermare, nelle acque internazionali, un natante privo di nazionalità sospettato di essere utilizzato per il trasporto illegale di immigrati e può ricondurre gli stranieri nel Paese dal quale sono partiti su richiesta del Paese cui appartiene, o si presume appartenga, l'unità navale. Questo è esattamente ciò che è avvenuto nei cosiddetti respingimenti nei confronti della Libia.

a queste operazioni. Ricordo, peraltro, che dall'agosto dell'anno scorso non si sono più verificati episodi di questo tipo, perché le autorità libiche hanno messo in atto un sistema di controllo delle coste, anche grazie alle sei motovedette che noi abbiamo consegnato loro, il che ha di fatto impedito la partenza di barconi di clandestini dalle coste libiche. quarto luogo, si chiede al Governo di mettere in atto politiche e programmi d'integrazione. Certamente, questa è una strada che il Governo ha seguito e continua a seguire. Quindi, prendo queste richieste come la conferma di un'azione un'azione che il Governo sta già svolgendo. Siccome sono abituato a parlare di fatti e non di chiacchiere, voglio solo citare la la dotazione finanziaria parziale delle iniziative che il Governo ha messo e mette in atto. Mi riferisco a quelle di competenza del mio Ministero,

in particolare nel programma-quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori 2007-2013» (programma europeo cosiddetto Solid), che conta un finanziamento complessivo di oltre 500 milioni di euro, suddivisi in quattro programmi: Fondo europeo per le frontiere esterne; Fondo europeo per i rifugiati, Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi e Fondo europeo per i rimpatri. Il primo, relativo alle

il quarto, per i rimpatri, conta 111 milioni di euro. Sono risorse già destinate in questi anni, secondo un programma che va dal 2007 al 2013, a finanziare una serie di progetti che vedono coinvolti gli enti locali, le Regioni, le Province

procedere anche speditamente sul fronte dell'integrazione, e non solo su quello della prevenzione degli ingressi clandestini. Anche su questo punto, quindi, le sollecitazioni nelle varie mozioni sono superflue, in quanto l'azione del Governo già si sviluppa in questa direzione. L'ultimo punto, su cui vorrei fare due considerazioni, è il rapporto con l'Unione europea. Si sollecita in molte delle mozioni un'azione del Governo italiano nei confronti dell'Unione europea. Sono iniziative che il Governo italiano ha già preso, e da tempo. Sin dall'inizio della mia azione di Ministro dell'interno ho chiesto, coinvolgendo anche i colleghi di altri Paesi del

Si fa spesso riferimento e si chiede spesso all'Italia di fare di più in materia di solidarietà. Ebbene, una volta tanto abbiamo chiesto noi ai Paesi europei di farlo, non solo con l'Italia, ma con quei Paesi situati sul confine del Mediterraneo e con i Paesi di primo ingresso dei clandestini. A noi tocca ricevere i clandestini che chiedono asilo e verificare se ci sono le condizioni e, una volta concessi i permessi di soggiorno per motivi umanitari, a noi tocca mantenere queste persone. Sono oltre 100.000 i rifugiati presenti in Italia. L'Italia registra tempi medi nettamente inferiori alla media europea per la valutazione delle domande di asilo (circa sei mesi contro i tre anni di media dell'Unione europea). Quindi, anche da questo punto di vista, l'Italia ha messo in atto un sistema tale da potersi considerare una *best practice* a livello europeo. Abbiamo chiesto ai Paesi europei ed alla Commissione di sviluppare azioni più incisive nella stipula di accordi bilaterali o multilaterali con i Paesi di origine, cosa che l'Unione europea non ha ancora fatto, ma comincia a ragionarci adesso. Abbiamo chiesto di potenziare la struttura di Frontex, cosa che l'Unione europea non ha fatto, ma comincia a fare ora, ed abbiamo chiesto di attuare il principio secondo cui, a prescindere dal Paese d'ingresso dei rifugiati, questi vengano collocati vengano collocati in tutti i Paesi europei per suddividere il peso (*burden sharing*) di questa collocazione. Di fronte a questa richiesta molti Paesi europei, in particolare quelli del Nord hanno detto: «No, grazie! Arrivano in Italia e ve li tenete voi». Credo che questo sia un principio che nega la solidarietà tra Stati membri. Ci siamo fatti carico e continueremo a farci carico comunque dei rifugiati, soprattutto dei minori. Su questo punto in particolare vorrei informare che l'Italia fa addirittura di più di quanto richiesto dalle normative europee: i minori che arrivano in Italia non vengono mai rimpatriati.

ma se sono minori noi li teniamo in Italia, non li rimandiamo in Grecia, pur potendolo farlo. Questo è un altro elemento che caratterizza le buone prassi italiane dal punto di vista dell'accoglienza e dell'integrazione, non solo del contrasto all'immigrazione clandestina.

là dove impegna il Governo a «cooperare con gli altri Paesi dell'Unione europea per un governo europeo dei fenomeni migratori,» - questa è la richiesta che il Governo italiano ha fatto fin dall'inizio della sua azione all'Europa - «affiancato da un nuovo modello di *governance*, che coinvolga tanto i Paesi d'origine, quanto quelli di destinazione dei flussi migratori, promuovendo intese e forme comuni di disciplina».

l'azione diplomatica che l'Italia svolge nel Mediterraneo è riconosciuta dai Paesi africani subsahariani e ha reso il nostro Paese il punto di riferimento di tutta l'Unione europea. a utilizzare a pieno gli strumenti della cooperazione allo sviluppo con i Paesi di origine e di transito, nella prospettiva di una più efficace *partnership* che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo»;

un esame più attento e più approfondito del suo contenuto avrebbe dovuto indurre il Ministro, a nome del Governo che rappresenta, ad esprimere un parere favorevole. Noi non siamo entrati nel merito della vicenda relativa al trattato con la Libia, né abbiamo espresso un giudizio di merito in proposito. Abbiamo rilevato che se le norme contenute nelle convenzioni internazionali e nella nostra Carta costituzionale che riguardano la garanzia del diritto d'asilo e della protezione umanitaria sono

del diritto di asilo e della protezione umanitaria e che ritenete prevalente rispetto alla tutela anche di un solo soggetto che ha diritto all'asilo, e alla protezione umanitaria un'operazione propagandistica sul modello sbarchi a Lampedusa. Ma vi state assumendo, signor Ministro, una responsabilità enorme, e non tanto per la politica interna di questo Paese, ma perché state delegando una materia che non potete delegare ad uno Stato estero. È vero in qualche modo riconosce la Convenzione di Ginevra, attraverso un complicato giro di norme e di convenzioni internazionali, ma se voi non affermate con i libici il principio in forza del quale il controllo anche presso i campi libici del rispetto di tali disposizioni è in capo al Governo italiano fate una cessione indebita di sovranità e vi rendete corresponsabili delle eventuali violazioni dei diritti umani che in quel territorio si svolgono, nell'ambito di una giurisdizione che è comunque dello Stato italiano. Questo è il punto.

a bordo delle navi (e qualcuno dovrà spiegarmi com'è possibile svolgere tali attività e conoscere se un soggetto vuole avvalersi della normativa sul diritto di asilo quando a bordo non c'è nemmeno un interprete che traduce: ma questo fa parte dei miracoli del vostro Governo),

donne incinta, persone che provengono dall'Eritrea e dalla Nigeria, cioè da Paesi in cui obiettivamente sono gravi problematiche per chi risiede, che mi sembra superfluo in questa sede dover rappresentare. Peraltro avrebbe dovuto farvi riflettere, signor Ministro, la circostanza che buona parte dei deportati di Rosarno

a mendicare in nero un lavoro nei campi perché il Governo non garantisce - non garantendolo gli enti locali che non hanno le necessarie disponibilità economiche - il becco di un euro

È allora chiaro che non ci meraviglia, signor Ministro, la sua dichiarazione; ci meraviglia il fatto che lei anche in questo caso non ha, secondo me, letto bene la risoluzione della Commissione affari esteri. Essa è molto ampia, molto complessa, tratta tutti i temi e afferma anche un principio in forza del quale non si può pensare che quando c'è un fallimento delle politiche sul contrasto all'immigrazione clandestina nel nostro Paese la responsabilità sia dell'Unione europea e quando, invece, avviene l'esatto opposto non vi sia alcuna responsabilità. Quindi, il problema va affrontato da molteplici visuali, senza ridurlo all'esaltazione all'esaltazione della norma sull'irregolarità o sul reato di immigrazione clandestina o delle altre disposizioni che poi hanno consentito ad alcuni sindaci del suo partito di fare operazioni tipo *White Christmas* (tanto per citare un esempio noto, ma ne possiamo citare tanti altri che riguardano amministratori leghisti, che, ad esempio, hanno problemi con il reato di istigazione all'odio razziale).

contratto di soggiorno, sul quale la Bossi-Fini è antecedente alla legge Biagi. Oggi una buona parte dell'irregolarità è quella che voi non contrastate, perché a voi non interessa contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina: a voi interessa semplicemente che sulle televisioni non si vedano gli sbarchi,

in equilibrio anche sotto il profilo dei conti previdenziali, deve avere una garanzia di immigrazione regolare annua di circa 300.000 unità; cifra che

a nessuno, neanche al Governo. Sul tema del mercato del lavoro è chiaro che una buona parte dell'irregolarità è determinata dalla rigidità dei contratti

aggravando la situazione di irregolarità che è determinata da quei contratti che hanno una durata molto breve e che riguardano anche i lavoratori extracomunitari, rispetto ai quali i flussi del mercato sono totalmente diversi da quelli immaginati dalla Bossi-Fini. Di tutto questo non volete discutere,

dalla legge comunitaria e che prevedeva sostanzialmente la riscrittura di tutte le norme in materia di mercato del lavoro, e di sfruttamento del lavoro nero, e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro extracomunitario. Tutti questi temi

questo provvedimento. Abbiamo presentato un disegno di legge *ad hoc* che si occupa di questo tema, ma non siete interessati a discuterne: a voi interessa solo agitare delle paure; a voi interessa solo fare una serie costante e stucchevole di *spot* elettorali, senza che a ciò corrisponda uno straccio di risultato concreto. Quando lei verrà qui, signor Ministro, e non ci parlerà di Lampedusa, ma ci parlerà di come il Governo ha ridotto il 90 per cento della immigrazione clandestina irregolare, che è determinata

sarà intrapresa, ad esempio, a Rosarno nei confronti di chi ha sfruttato il lavoro nero degli extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, allora avrete la credibilità per affrontare seriamente questo problema. Ad oggi, la sua relazione è solo deludente e noi non possiamo che votare contro la mozione presentata dal

confesso di essere rimasto abbastanza deluso dall'approccio che il Ministro dell'interno ha manifestato nell'affrontare l'atto che quest'Aula sta esaminando (ossia l'atto comunitario n. 17), la risoluzione approvata all'unanimità comunicata alla Presidenza il 15 aprile 2009 e, ancora più importante, la relazione

Eppure questi documenti dovevano costituire uno stimolo importante per una discussione che è mancata nel Parlamento. lei ci ha rassegnato una serie di numeri, ma il limite culturale all'approccio del problema è troppo manifesto. L'atto comunitario n. 17 individua la necessità di un approccio globale al problema e testualmente afferma: «L'approccio globale riflette la profonda trasformazione subita negli ultimi anni dalla dimensione esterna della politica di migrazione europea: da un'impostazione incentrata principalmente sulla sicurezza e focalizzata sulla riduzione delle pressioni migratorie si è passati a un approccio più trasparente ed equilibrato, guidato da una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno e volta a migliorare le misure di accompagnamento e di gestione dei flussi migratori, per trasformare migrazione e mobilità in forze positive a favore dello sviluppo». di una sollecitazione ad affrontare un problema che ha caratterizzato l'esordio di questo Governo. Forse se quest'atto e questa risoluzione avessero preceduto le iniziative legislative di questo Governo all'inizio della legislatura, gli esiti sarebbero stati diversi,

di immigrati nel nostro Paese produce il 9,6 per cento del prodotto interno lordo nazionale. L'Europa sta invecchiando e questo è un dato che viene offerto alla nostra valutazione:

Secondo gli studi delle Nazioni Unite, nel 2050 entreranno nel mondo del lavoro 438 milioni di uomini e donne provenienti per il 97 per cento da Paesi in via di sviluppo. Su questi dati dobbiamo impostare la nostra lettura, non sulla rassegna di quanti immigrati in meno sono sbarcati sulle nostre coste. Dobbiamo confrontarci con un fenomeno che non bloccheremo, perché è mondiale e globale, con il reato di ingresso e soggiorno illegale nel nostro Paese, punito con l'ammenda sino a 5.000 euro, come se il il migrante che sbarca sulle nostre coste abbia la carta di credito per pagare l'ammenda, sapendo che qualora non la paghi - non la pagherà - l'alternativa è quella di sostituire la pena dell'ammenda con l'obbligo di risiedere nel proprio domicilio nei giorni di sabato e domenica; questo stabilisce la legge, cioè una cosa ridicola. La risposta muscolare che il nostro Paese Paese sta dando non tiene conto della globalità e dell'imponenza del problema, che rappresenta una sfida per i prossimi anni. Ma veramente pensiamo di affrontare i problemi in termini di sanzioni, con quest'assurda invenzione dell'aggravante della clandestinità per qualunque reato commesso? Una violazione qualunque, anche al codice della strada, un incidente stradale è punito più gravemente se l'ha commesso un clandestino rispetto al cittadino italiano o europeo. C'è questa assurda aggravante inventata, così come il problema del reato di immigrazione e di soggiorno illegale. L'Europa ci dice - e la risoluzione che noi qui approviamo e che lei ha condiviso lo afferma, ma evidentemente ha prestato poca attenzione - che, che, concentrandosi sugli aspetti più immediati e controversi dell'immigrazione, si accentua la percezione negativa e frequentemente la politica, invece di sedare, cavalca la paura in cambio di facili consensi; nascono così risposte di corto respiro che, se placano per qualche giorno i cittadini, molto spesso generano incertezza e confusione. Questo è ciò che dovevamo discutere, così come come dobbiamo apprezzare la profondità e l'alta visione che la risoluzione, accompagnata dalla relazione del presidente Pisanu, ci hanno offerto come materia di discussione, laddove si dice l'immigrazione è una necessità storica ed è la sola concreta alternativa alla decadenza. Allora dobbiamo denunziare il fatto che la vostra concezione, e anche la sua, signor Ministro, risponde a un approccio superato, antico, non più adeguato alla realtà. Come si dice nella risoluzione, che pure lei approva, fino a ieri, pur traendone enormi benefici, l'Europa ha percepito l'immigrazione in maniera negativa e pertanto ha adottato politiche sostanzialmente difensive, rivolte cioè a contrastare l'immigrazione clandestina ed a limitare Oggi c'è un'altra impostazione mondiale sul problema e, purtroppo, l'occasione che ci era stata offerta da questa importante risoluzione, accompagnata dalla relazione del presidente Pisanu, non ci è servita per affrontare seriamente - al di là dei numeri, del conto della spesa che lei ci ha presentato - e non ha per nulla sfiorato la grande sfida che siamo costretti ad affrontare e che dovremo affrontare nei prossimi anni; nessuna parola in questa direzione. Noi invece vogliamo confrontarci sul problema con un discorso alto, impegnativo, e non di corto respiro per dare risposte mediatiche alle esigenze momentanee e ai timori

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, innanzitutto il Gruppo della Lega Nord voterà a favore della risoluzione presentata dalla 3a Commissione permanente perché ne condivide il dispositivo, il dispositivo, il quale contiene un impegno che possiamo tranquillamente sottoscrivere. Non condivide alcuni passaggi della relazione del relatore, collega Pisanu, soprattutto quelli che alcuni colleghi dell'opposizione hanno richiamato in senso entusiastico, laddove - per esempio - si dice che nei prossimi vent'anni l'Italia avrà bisogno mediamente di 300.000 nuovi immigrati all'anno. Noi abbiamo gli occhi e vediamo una situazione del mercato del lavoro totalmente in difficoltà in questo Paese. Non possiamo quindi pensare che detto contingente numerico di 300.000 immigrati all'anno possa essere un parametro realistico e - come dire - anche intelligente. di una affermazione ovviamente di carattere ideologico e priva di ogni supporto di verifica concreta dei dati dell'attuale situazione del mercato del lavoro.

questo il principio cardine ed il motivo per il quale non possiamo condividere alcune affermazioni, come quella che ho prima citato, della relazione Pisanu. Peraltro, in detta relazione sono contenuti anche alcuni passaggi che ci convincono, come - per esempio - quello secondo cui l'immigrazione clandestina va combattuta; è una patologia grave, perché ha una forte incidenza sull'andamento della delittuosità complessiva. Finalmente, anche in una relazione

sentito negare l'evidenza di tale correlazione. Ovviamente, accanto al voto favorevole alla nostra mozione, ne esprimeremo un altro favorevole alla mozione presentata dal Gruppo del Popolo delle libertà, anche se - come ha sottolineato correttamente il ministro Maroni non sono ammesse regolarizzazioni o sanatorie generalizzate, essendo vietate dal Patto europeo sulla immigrazione e l'asilo. Quindi, qualsiasi riferimento a regolarizzazioni non può riguardare le sanatorie generalizzate, bensì - come dice il Patto europeo sull'immigrazione e asilo - regolarizzazioni caso per caso, che vuol dire proprio persona per persona, laddove ci siano le condizioni e i requisiti che la stessa legge Bossi-Fini prevede in diversi suoi articoli. con una semplice affermazione. L'unico Paese europeo che, al di là del luogo comune dell'immigrazione come risorsa, ha fatto una indagine econometrica sui costi e i benefici della stessa,

contenuto in una relazione molto precisa nella sua valutazione e nei suoi dati anche economici. Il risultato quindi è una sconfessione di quel luogo comune, di cui spesso sentiamo riempirsi la bocca alcuni esponenti dell'opposizione, secondo cui l'immigrazione è una risorsa. Valutiamo anche noi, come ha fatto l'Inghilterra, se davvero si tratta di un luogo comune o se corrisponde alla realtà dei fatti. In Inghilterra lo hanno fatto e hanno visto che era un luogo comune e che in realtà i fatti dimostravano esattamente il contrario, e per questo hanno cambiato le politiche sull'immigrazione. Stanno studiando - ormai è quasi in fase di entrata in vigore - una politica selettiva dell'immigrazione basata su un sistema a punti dove si va ad individuare l'immigrato in funzione delle caratteristiche professionali e del titolo di studio che possiede. Si sceglie così un'immigrazione qualificata e non portatrice di problemi sociali (così la definisce l'*House of Lords* nel suo rapporto). Credo che abbiamo iniziato anche noi un percorso verso la direzione di un'immigrazione più qualificata e più controllata. È la direzione giusta, e proseguiamo così.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Partito Democratico ho l'onore di dichiarare il voto a favore del provvedimento in esame per le ragioni esposte nella limpida e argomentata relazione del senatore Pisanu. In essa fa spicco l'esigenza, definita "di fondo", di affrontare il tema dell'integrazione di migliaia e migliaia di immigrati nel nostro tessuto economico e sociale. E' qui che, nella consapevolezza di quanto il compito sia arduo, l'azione politica eleva anche a dimensione morale uno dei più complessi e controversi problemi di cui sia stato investito il Parlamento della Repubblica. In tale impegno si concreta il riconoscimento ai migranti nel nostro Paese del medesimo rispetto che dobbiamo a noi stessi. E' il senso più profondo della democrazia: la pari dignità legata ai diritti che la Costituzione riconosce e garantisce. Ciò di cui ci occupiamo cade in un tempo nel quale occorre convincersi che ciascuna delle nostre culture, delle nostre fedi, delle nostre costruzioni sociali, delle nostre conquiste civili ha per destino d'implicarne altre che già interpellano la nostra autenticità democratica, i nostri principi, la nostra etica. "Il tempo della reciprocità - avvertì lo storico Fernand Braudel - è più che alle porte". Non ascoltammo, o non abbastanza. Soltanto oggi, quando la questione si è fatta grave, abbiamo capito che opporvisi è accettare la divisione, lo scontro, la perdita della comunanza. Che cosa, allora, è ragionevole fare? Osservare le leggi, prima di tutto. Ma a condizione che siano buone leggi, cioè accompagnate non solo dalla loro certezza normativa, ma anche dalla percezione dell'"altro", del suo stato, della sua sopravvivenza, nella consapevolezza che gli uomini non solo "esistono", ma "vivono" insieme. Di fronte a quanti soccombono - perché vittime della loro storia - un laico d'ingegno e di cuore si lanciò in questo bellissimo azzardo: «*Pietas*, prima luce della giustizia!». Si chiamava Gaetano Salvemini, storico, politico, umanista del nascente socialismo italiano. Lo stesso che, in un'altra circostanza, ebbe a dire che «parlare di razza è un'assurdità, perché è la Storia a determinare l'identità dei popoli». In materia di giustizia non pronunciò parole diverse il compianto direttore della Caritas romana, don Di Liegro, animatore di un fronte umanitario istituito per la difesa degli altri, i deboli, gli attardati e, appunto, i soccombenti. Lo intervistai a lungo scoprendo che si può essere caritativi, e al tempo stesso solidali, quando si sappia praticare, senza venir meno al proprio dettato interiore, la distinzione tra il verbo redimere e il verbo liberare. «Gli economisti» - mi disse - «affermano che l'orizzonte temporale delle scelte si è di molto accorciato: s'investe poco sul futuro, non si guarda abbastanza oltre la propria capacità di accumulare e disperdere. La storia di questi ultimi anni è stata un grande, pantagruelico banchetto in cui i commensali hanno divorato tutto il possibile, senza badare a chi sarebbe venuto dopo. Solidarietà - aggiunse - è anzitutto legalità. Essere solidali con gli emarginati implica lo sforzo di sentirsi simili a loro. Altrimenti è il rifiuto, a priori, della giustizia». Pesa sulla nostra coscienza la povertà di quei popoli cui abbiamo chiesto addirittura il pagamento degli interessi su ciò che avevano ricevuto perché non ci disturbassero durante lo sfruttamento delle loro risorse. È ora di cominciare a credere che nell'epoca dell'abbondanza si muore di fame più di quanto non accadesse ai tempi della miseria endemica. Dopo anni dall'impegno a diminuire la fame nel mondo, 854 milioni di persone non hanno cibo a sufficienza: il numero degli affamati è cresciuto. Oggi, per paradosso, i poveri sono più indifesi rispetto a quando un mondo prevalentemente contadino dovette gestire una «civiltà del meno», chiamata anche della sopravvivenza. Allora si diffuse una sorta di regola che fece della miseria generalizzata una struttura della vita quotidiana, secondo una diagnosi realistica di quei tempi. Altra cosa è la povertà di oggi, quando nessuno strumento empirico e utilizzabile mondialmente è in grado di ridurre e, in un certo senso, calmierare la fame. Il villaggio dell'abusato McLuhan, credetemi, non è globale. Nel Sud della terra muoiono ogni giorno di fame, inedia e malattia circa 30.000 bambini: circa 500 *jumbo* stipati di bambini ogni giorno precipitassero sulla crosta terrestre. Ditemi se non avremmo motivo di celebrare tutte le sere una sorta di lutto universale. C'è di più: a poco più di 200 anni dalla nascita dei "lumi", almeno un miliardo di persone non conosce ancora la luce elettrica. Vengono così abbandonati, all'inedia, alla rassegnazione e alla resa moltitudini di «attardati», una specie di lascito fisiologico della storia, secondo una gelida diagnosi del pragmatismo economico non ancora sbugiardata del tutto. Per l'avvenire dovremo disporci a una ponderata accoglienza in ragione di un'adeguata cittadinanza, senza venir meno all'impegno di favorire la crescita dei Paesi da cui gli immigrati provengono; altrimenti, la semplice forza del numero prima o poi sarà destinata a sommergerci e ciò accadrà quando i poveri si saranno definitivamente stancati di essere soltanto e per sempre i poveri. Se non saremo pronti, sarà la demografia a decidere la partita, cioè a governare un processo che la politica e l'etica avrebbero dovuto guidare. Non userò, per mera bonomia intellettuale, il ragionamento secondo cui, vivendo in una società multi-etica, essa ci trasformerà, l'un l'altro, in una sorta di «stranieri morali»; il che postula, *a priori*, il concetto e poi la pratica della tolleranza e della solidarietà. Domandiamoci piuttosto se non dipenderà da tutti noi affrontare il problema costituito da un mondo dove il 52 per cento dell'umanità è povero; il 38 per cento si divide tra il viver bene e il disporre del necessario e il 10 per cento è più ricco di tutto il resto messo insieme. Abbiamo alle spalle un Novecento colpevole di tanti orrori, ma al qual va riconosciuta la più civile e morale delle scoperte antropologiche: il valore del "noi" valutato in rapporto a quello, pur prezioso, dell'io. Oggi, permettetemi l'immagine, stiamo rimettendo sui telai quella tela solo apparentemente astratta che è la storia delle nostre scelte profonde, civili e morali, per dirla con Goethe. Il testo che voteremo è un invito a guardare questa Aula come a un luogo in cui è possibile rimettere insieme le ragioni per le quali siamo qui a parlare in nome della nostra civiltà, cioè del nostro voler essere per la giustizia con l'orgoglio e la responsabilità, signor Ministro, di renderla viva e operante. Siamo qui a dirci, non a declamare, che la Storia siamo noi a condizione di non esserlo a scapito di chi, non per sua colpa, ne ha conosciuto fin qui solo un simulacro. *(Vivi

oggi pomeriggio in questa Aula parte da un punto di profonda verità che noi non possiamo non condividere.

con coscienza, affermare essere la ricetta vincente. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo legato a tempi nuovi. La vecchia immigrazione, quella novecentesca, era prevalentemente legata a fenomeni di tipo coloniale e questa sua origine era fondamentale nella definizione dei modelli, delle ricette con le quali i grandi Stati colonialisti, i grandi imperi, hanno gestito il fenomeno. In sostanza, due sono stati i modelli che si sono stagliati nel nostro Novecento. Il primo fu l'assimilazionismo francese, quello per cui l'immigrato era sottoposto ad una sorta di religione di Stato del Paese ospitante, che lo assorbiva e che gli consentiva di diventare cittadino di quello Stato dopo un certo numero di anni. Era il modello fondato sulla centralità della scuola pubblica intesa come tempio del sapere laico nel quale il maestro tramandava le tavole della cittadinanza di generazione in generazione. è il motivo per il quale la scuola in Francia, anche dal punto di vista architettonico, è stata immaginata quasi come un tempio; il motivo per il quale la polemica tra scuola pubblica e scuola privata in Francia ha assunto una centralità che non ha avuto in nessun altro contesto del continente europeo. Ma quel modello, che si rifaceva alla geopolitica del Novecento, è fallito sotto i nostri occhi.

di culture che si giustapponevano alla cultura della comunità accanto trovando dei princìpi di legittimità interna, condizionando in questo modo la legittimità unificante del riferimento statuale.

messo in dubbio dagli attentati che si sono verificati nelle metropolitane di Londra da parte di

il multiculturalismo con il suo nome: un incubo dal quale sfuggire per ritrovare punti di riferimento più sicuri, per ritrovare sintesi culturali più stabili a dispetto delle dimensioni che il fenomeno dell'immigrazione stava assumendo. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno, quello dell'età della globalizzazione e del nuovo secolo, che non ha paragoni con quello del secolo che abbiamo alle spalle. È cambiata completamente la geopolitica dell'immigrazione, creando problemi, tra l'altro, a Paesi come il nostro che, dal punto di vista geopolitico e delle frontiere, si trovano particolarmente esposti. È cambiata la permeabilità delle frontiere che prima erano superabili con molta più difficoltà di oggi. Non a caso i sociologi del fenomeno dell'immigrazione hanno coniato formule fino a poco tempo fa sconosciute: siamo venuti a conoscenza della circolarità del fenomeno dell'immigrazione, che non si ferma più in un Paese, ma che spesso si muove da un contesto all'altro, come della sua temporaneità: un tempo, come si diceva nelle canzoni popolari, quando si prendeva la nave per andare dall'altra parte dell'oceano si riteneva di non tornare più a casa o lo si faceva in due o tre occasioni spesso l'immigrato non perde il rapporto con il luogo di origine, ma anela a tornarvi dopo un periodo di permanenza in un'altra terra o molto spesso in altre terre. Sono questi motivi che devono portare anche a un ripensamento profondo del rapporto che esiste tra l'immigrazione, l'integrazione e la cittadinanza: sono tre categorie e tre problemi differenti. Sovrapporli come fossero la stessa cosa sarebbe un grave errore: non un guardare indietro, ma un guardare da un'altra parte rispetto alle caratteristiche che il fenomeno ha assunto oggi. oggi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se questa è la situazione nuova di un fenomeno nuovo è inutile riproporre le vecchie logiche e le vecchie contrapposizioni tra rigore e buonismo. È inutile tornare tornare alle vecchie categorie. Dobbiamo ammettere che ci troviamo su un terrenodi sperimentazione nel quale molto c'è da trovare e pochi sono i punti di riferimento certi che abbiamo. Per quel che ci riguarda alcuni li vogliamo indicare e li abbiamo inseriti nella nostra mozione: innanzitutto, il rispetto del principio la soluzione del problema, ma è un punto di riferimento dal quale non si può prescindere nella ricerca di un nuova strategia e di una nuova politica. Vi è poi la considerazione, accanto alle debolezze tradizionali, delle nuove debolezze che sono legate anche alla novità del fenomeno. Signor Presidente, noi soltanto la debolezza degli immigrati che arrivano nel nostro Paese e che molto spesso sono spinti dalla disperazione e dalla ricerca di una vita migliore. C'è anche la debolezza di parte dei nostri cittadini che subiscono le conseguenze di un fenomeno fuori controllo. Dobbiamo guardare a cosa accade nelle *banlieue* delle grandi città italiane. Dobbiamo considerare le nuove paure che si instaurano e che sono spesso altrettanto ingiuste della condizione di quanti arrivano qui cercando una vita migliore. Inoltre, dobbiamo essere accorti tutelare i diritti fondamentali di quanti arrivano nel nostro Paese, perché non basta ospitarli. È uscita oggi una bellissima pubblicazione di una parlamentare del Popolo della Libertà, Souad Sbai, nella quale si racconta nel dettaglio quali siano le debolezze delle donne immigrate che non vengono tutelate dalle nostre leggi nelle loro comunità di origine. Non possiamo girare la testa dall'altra parte e mondarci la coscienza senza guardare a questi autentici drammi, come sono drammatiche le condizioni dei bambini vengono ridotti in regime di semischiavitù ancor peggio che nei loro Paesi di origine. Queste nuove debolezze vanno considerate insieme alle vecchie nella ricerca di punti di caduta che non sono affatto scontati. È questo quello che deve muoverci e che deve portarci a modulare quantità e qualità nell'accoglienza agli immigrati nel nostro Paese. L'ultimo punto di riferimento che vorrei

le culture siano mobili, che le culture cambino, che siano in movimento e che si integrino continuamente, a differenza delle religioni, soprattutto quelle rivelate, che fanno riferimento a dogmi e che, in quanto tali, non si possono mettere in discussione. Non è questo il problema; e rivendicare un'identità non vuol dire essere, o battersi, per una cultura che rimanga immobile. Vuol dire

Sulle radici cristiane si è giocata una partita che è andata al di là del problema puramente nominale. Il problema è se la nostra identità debba essere determinata anche da quello che siamo stati e dalla responsabilità che ciò implica possa essere intesa solamente come qualcosa in divenire, che si deve formare sulla base di diritti che producono continuamente nuovi diritti, facendoci dimenticare cosa siamo stati e da dove proveniamo. *(Applausi dal che abbiamo di fronte. È la battaglia tra una libertà intesa soprattutto come responsabilità e una libertà intesa soprattutto come diritto che produce sempre diritti nuovi, nell'illusione che, in questo modo, la persona possa essere effettivamente più libera, e non più sola perché priva anche di quei riferimenti che costituiscono le sue radici.

hanno determinato un mutamento del ruolo dello Stato e hanno messo in evidenza anche il cambiamento dei suoi compiti, mostrando anche come lo Stato non possa più assolvere alcune sue funzioni novecentesche e dovrà assolverne altre estremamente più importanti; e, a fronte di questa realtà, fino ad oggi su questo fenomeno l'approccio è stato prevalentemente statalista. Ogni Stato ha cercato di scaricare sul vicino gli oneri di questo di questo grande problema. Ricercare un approccio comunitario e solidale è la via giusta, senza dimenticare quei punti fissi che sono l'unica bussola che deve guidarci in una ricerca verso il nuovo.

n. 16, approvato dalla 3a Commissione permanente, in linea con una prassi consolidata, le connesse mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

**Il Senato non approva.**

con tutto lo sdegno possibile e comprensibile le dichiarazioni platealmente offensive e provocatorie del presidente Gasparri in relazione a presunti brogli elettorali in Australia di cui io sarei il beneficiario. Sfido il presidente Gasparri o chiunque a trovare, a portare un solo atomo di prova circa quanto ha riferito sulla scorta di un articolo diffamatorio del quotidiano «Avvenire», e solo di quel giornale, contro il quale è stata già sporta denuncia per diffamazione da parte mia e del collega, anche eletto in Australia, della Camera dei deputati, onorevole Marco Fedi. Ad informazione del presidente Gasparri, io sono stato onorevolmente ed ampiamente eletto, rieletto e confermato in Australia e nel resto della circoscrizione Oceania, Asia ed Africa in maniera totalmente trasparente, infinitamente più pulita di vari colleghi del partito del presidente Gasparri, incluso quello di cui ci stiamo interessando in queste ore. In questa occasione, per ragioni che conosco bene e sulle quali non intendo dilungarmi ora, perché sono in corso azioni giudiziarie nel nel foro di Roma e in Australia, il già austero organo della CEI si è trasformato in organetto da straccioni e farabutti con licenza di vilipendio, ma nessuno può consentire al collega Gasparri, in quest'Aula, altrettanta licenza di vilipendio. Quanto ha dichiarato, per la sostanza e per la forma in cui l'ha fatto, può essere interpretato come frutto di disonestà intellettuale, che non fa onore né a lui, né al suo Gruppo, né a questa Assemblea. Il tuo abituale bullismo, collega Gasparri, non mi impressiona!

si trova in liquidazione a seguito del crack del precedente proprietario, il quale l'aveva acquisita in amministrazione controllata.

erano state addirittura staccate le utenze. Ma, a seguito dell'intervento delle istituzioni locali (il Comune e la Provincia), oggi si è ripristinata la capacità produttiva dell'azienda.

In questo momento, e fino ad oggi, l'atteggiamento dei lavoratori è stato ed è corretto, ma sappiamo bene come il timore della perdita del posto di lavoro dopo giorni di tensione possa anche riscaldare gli animi. Chiedo quindi al Governo di attivarsi in tutti i modi per verificare velocemente quale sia la reale situazione, che rischia di precipitare nelle prossime ore, e di attivare tutti gli strumenti necessari a disposizione per recuperare una proficua ripresa della normalità delle relazioni economiche e sociali di quella comunità.

Signor Presidente, è ancora viva e forte l'emozione per il terremoto che ha colpito Haiti per il quale si è subito avviata tutta l'azione di sostegno e di solidarietà internazionale), che è avvenuto un altro grave evento naturale, il terremoto che ha colpito un Paese del Sud America: il Cile.

Oltre alla cassa integrazione e, ora, alla chiusura di questa azienda, vi è forte preoccupazione per il degrado ambientale in in cui versa il suo stabilimento. Vi sono gravi contaminazioni da amianto che mettono in pericolo una vasta area geografica; praticamente non è un problema meno grave di quello che si è verificato a Casale Monferrato. Ora, sembra che sia stato annunciato dal sottosegretario Letta, alcune settimane fa, un intervento immediato di bonifica mediante l'inserimento dell'intero complesso tra i siti di bonifica di interesse nazionale.